Onorevoli colleghi, un nostro militare, l'alpino caporal maggiore Giorgio Langella, è caduto oggi in un attentato a Kabul e altri cinque soldati, anche loro alpini, sono rimasti feriti; due, in modo particolarmente grave. Si tratta di un ulteriore, pesante tributo che l'esercito italiano paga alla causa della pace. A nome dell'intera Assemblea del Senato e mio personale, esprimo i sentimenti di commosso cordoglio e di solidarietà alla famiglia del caporal maggiore Giorgio Langella e formulo l'augurio di un pronto e completo ristabilimento ai militari feriti. Per onorare la memoria del soldato rimasto vittima nell'adempimento del proprio dovere, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

Signor Presidente, mi associo alle sue parole. Vorrei esprimere a nome mio personale, e credo di tutta l'Assemblea, i sentimenti di una profonda e condivisa partecipazione al dolore dei familiari del caporal maggiore Giorgio Langella, rimasto vittima di un vile attentato a Kabul. L'ennesimo sacrificio di un giovane impegnato nel nome del proprio Paese in una missione militare difficile, in un'area devastata da conflitti interetnici. Mi sento intimamente vicina alla famiglia perché conosco quel profondo dolore che si prova davanti a una vita spezzata, a un futuro incompiuto, al vuoto che lascia la scomparsa di una persona cara, cara anche a tutti noi. Un pensiero affettuoso e un augurio vanno anche al caporal maggiore Salvatore Coppola, al caporale Sebastiano Belfiore e al caporale Pamela Rendina, rimasti feriti nell'agguato, nonché alle vittime civili e a quella tenera vita distrutta. Ai nostri militari esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra gratitudine per il loro contributo, teso a costruire uno scenario di pace in un teatro che permane ostile. Altrettanto ci colpisce e ci addolora, per la sua efferatezza, l'assassinio di Safiya Amajan, responsabile delle questioni femminili della provincia di Kandahar, che svolgeva, con impegno e passione, il suo lavoro per garantire alle donne dell'Afghanistan pari diritti e opportunità ed un ruolo nel futuro del proprio Paese.

*dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia:* «Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche» Onorevoli colleghi, nella giornata di mercoledì 27 settembre 2006 avranno luogo le sedute costitutive delle delegazioni italiane presso le Assemblee parlamentari dell'UEO, del Consiglio d'Europa e della NATO. Per le ore 14 è convocata, presso la Camera dei deputati, sede di Vicolo Valdina, la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Unione

Per le ore 15 è convocata, presso l'Aula della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica, la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO. Porto a conoscenza dell'Assemblea che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha adottato all'unanimità modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 5 ottobre. La discussione generale sul disegno di legge recante sospensione dell'efficacia di disposizioni dell'ordinamento giudiziario proseguirà oggi pomeriggio fino alla conclusione degli interventi. La seduta potrà pertanto protrarsi, a tal fine, fino alle ore 22. Le repliche del relatore e del Governo saranno svolte in apertura della seduta antimeridiana di domani. Avrà quindi inizio la fase delle votazioni, con la trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti. Le votazioni potranno proseguire fino a tutta la seduta antimeridiana di giovedì 28 settembre, con eventuale prolungamento fino alle ore 15, ove necessario alla conclusione dei voti sugli emendamenti. In ogni caso, le dichiarazioni di voto e il voto finale avranno luogo nella seduta pomeridiana di martedì 3 ottobre. Nella seduta antimeridiana dello stesso giorno saranno discussi il bilancio interno e il rendiconto del Senato. I relativi ordini del giorno dovranno essere presentati entro le ore 19 di domani, mercoledì 27 settembre. Il calendario prevede poi l'esame dei disegni di legge e dei documenti relativi alle Commissioni d'inchiesta su mafia, rifiuti, infortuni sul lavoro e uranio impoverito, nonché, se concluso dalla Commissione competente, del decreto-legge in materia di detraibilità dell'IVA. Nella seduta antimeridiana di giovedì 5 ottobre, alle ore 9, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni al Senato sulla vicenda Telecom. Modalità e tempi del dibattito saranno definiti dalla prossima Conferenza dei Capigruppo. In tale riunione sarà anche stabilito in quale seduta, compresa tra il 10 e il 12 ottobre, saranno poste all'ordine del giorno mozioni sulle vicende connesse al discorso tenuto da Papa Benedetto XVI a Ratisbona.

È iscritto a parlare il senatore Mantovano. Ne ha facoltà.

ma io mi specchio nelle spalle del senatore Russo Spena, che è persona garbatissima. dei temi trattati e ci fu risposto che, nel corso dei lavori parlamentari, si sarebbero avviate tutte le iniziative opportune per riempire di contenuti l'esigenza fortemente avvertita di cambiare alcuni segmenti importanti della giustizia. Devo dire che l'unica iniziativa sulla quale la maggioranza si sta spendendo, con un vigore che forse - anzi senza forse

Signor Presidente, capisco che i temi trattati, quando si parla di argomenti triti e ritriti, non appassionino più di tanto.

che sta creando in alcuni settori del Paese, peraltro non secondari, forti conflitti. Parlo di forti conflitti perché trovo francamente singolare, signor Presidente, che l'attuale maggioranza abbia fatto proprie indicazioni che venivano da un'importante associazione di categoria, l'Associazione nazionale magistrati, e in forza di questi *input* - e soltanto in forza di essi - abbia proposto questo disegno di legge, teso a sospendere l'efficacia della legge che noi approvammo, dopo un lungo e complesso *iter*, nella scorsa legislatura. legge che venne sottoposta al vaglio della Presidenza della Repubblica, la quale pretese giustamente taluni cambiamenti e modificazioni che furono apportate, di talché il prodotto finito appariva certamente congruo e conferente rispetto alle esigenze di modernizzazione da tutti avvertite. Non posso, signor Presidente, non tornare su un tema già trattato nel corso della discussione sulla questione pregiudiziale: a quali regole si dovrà uniformare la magistratura nel momento in cui dovesse essere sospesa,

trovo singolare che si possa evocare, da parte della maggioranza, l'articolo 97 della Costituzione a sostegno dell'inconferenza dell'apparato normativo di cui oggi si chiede la sospensione, considerando che poi si dovrebbe affrontare, per un certo periodo di tempo, certamente non secondario, una *vacatio legis* assolutamente ingiustificata.

quale legge sarà applicata fino al luglio 2007? Pongo tale interrogativo all'Aula e rimarco l'importanza di questo argomento, perché ritengo che questo tema non potrà non essere rassegnato alle valutazioni della Corte costituzionale.

perché è proprio sulla parola che ha improntato le ragioni del suo essere e ancora coltivo l'illusione che le parole possano essere disapprovate o apprezzate, ma debbono comunque essere valutate.

la mia resta un'aspirazione. Voglio sperare che non sia così, signor Presidente. Signor Presidente, perché abbiamo bisogno di una magistratura altamente professionale? Perché abbiamo bisogno di una magistratura capace, di una magistratura rigorosa, di una magistratura che abbia piena consapevolezza del proprio ruolo? Io dico: perché i limiti della politica hanno imposto questo sistematico controllo di legittimità. Sono perfettamente edotto che questa transizione, che non si è conclusa,

Ogni giorno leggiamo di ineffabili realtà che si scontrano e che impongono il rigoroso controllo di legittimità della magistratura. Qual è allora la conseguenza? Se io ammetto - e non posso fare diversamente, perché questa è la situazione - l'importanza della funzione, debbo pretendere che la funzione stessa sia esercitata con il massimo rigore. Debbo avere la piena consapevolezza e la piena cognizione che i soggetti cui è demandata questa funzione così importante,e così fortemente incidente sulle realtà che riguardano altri uomini siano tutti soggetti particolarmente qualificati e a questo fine, signor Presidente, onorevoli colleghi, tendeva

Una dialettica che cominciò fin dall'inizio, quando trattammo questi temi sensibili, non solo con l'opposizione dell'epoca, ma anche con l'Associazione nazionale magistrati. Rammento la costituzione di tavoli di concertazione, nel cui ambito si discussero questi argomenti e si immaginarono soluzioni condivise; tutto ciò finché non irruppe lo sciopero dei magistrati, che certamente pose termine a quel dialogo altamente produttivo. La disponibilità a trattare, signor Presidente, non è venuta meno nemmeno adesso. Noi difendiamo con grande determinazione la legge che nella scorsa legislatura fu promulgata, però non siamo insensibili alla possibilità di sedersi ad un tavolo di lavoro ed immaginare delle soluzioni. Perché questaiattanza da parte del Governo e della maggioranza di chiedere la sospensione? Una iattanza che poi confligge, signor Presidente, con gli argomenti che sono stati trattati dal Ministro Guardasigilli, perché quest'ultimo ha esposto, in una compiuta relazione, tutta una serie di ipotesi alternative che avrebbero potuto formare oggetto di un disegno di legge sul quale discutere. Perché dobbiamo differire di qui a luglio la trattazione di questi temi e non discuterli adesso? Trovo confliggente, signor Presidente, questo atteggiamento del Governo, lo trovo francamente illogico: da una parte sospendo e dall'altra propongo. Non voglio usare le espressioni che nella scorsa legislatura venivano adottate sistematicamente per definire l'attuale legge, di cui allora discutevamo, controriforma, per l'amor del cielo. di un problema di controriforma. Vi sono esigenze che possono essere prese in considerazione, ma

scelte. Signor Presidente, quando viene evocato in maniera enfatica

francamente resto perplesso. Trovo veramente singolare che non si sia immaginato - perché lo si è immaginato e lo si applica - il sistema della cosiddetta archiviazione per pacchi.

nei sistemi giudiziari e permetterebbe di risolvere una serie di vicende che non andrebbero certamente ad appesantire in alcun modo le attività più impegnative che, sotto questo profilo, il Consiglio potrebbe realizzare. signor Presidente, che l'aspirazione più avvertita nel Paese in tema di disciplina sarebbe un'altra e mi sarebbe piaciuto che l'attuale maggioranza,

immaginando la soluzione auspicata di un organismo autonomo rispetto al Consiglio superiore che si possa occupare esclusivamente di disciplina.

ciò che dichiararono alcuni autorevoli esponenti, vertici dell'Associazione nazionale magistrati, qualche tempo fa, proprio a proposito della disciplina, quando sostennero

Allora, se questa è la ragione che imponeva un intervento e siccome non viene proposto un intervento radicale e fortemente avvertito,

singolare che invece di discutere di questi argomenti, invece di dare un contributo al cambiamento e al miglioramento, si voglia sospendere correndo il rischio di non realizzare alcunché e di ricadere poi nella situazione che adesso si intende tenere per un attimo in un angolo. angolo. Signor Presidente, un altro aspetto che ha suscitato grandi critiche da parte di osservatori superficiali - me lo consenta - è stato quello afferente il cosiddetto concorsificio, un'espressione pittoresca

l'attitudine, il rigore di chi poi deve realizzare progressioni di carriera; soluzione che si contrappone naturalmente a quell'automatismo che da tempo è stato denunciato da ogni parte politica, salvo poi modificare l'atteggiamento nel momento in cui le contingenze imponevano le contrapposizioni. Tutti hanno lamentato atteggiamenti di questo genere. Ebbene, rispetto a questo profilo della norma, della quale oggi voi chiedete la sospensione, cari colleghi della maggioranza, noi manifestammo disponibilità massima alla trattazione. Dicemmo che l'ipotesi di riconsiderare questo aspetto ci vedeva, tutto sommato, disponibili: lo dicemmo in sede di Commissione, lo abbiamo detto nei convegni e in mille colloqui che abbiamo tenuto sull'argomento. L'unica cosa alla quale tenevamo e teniamo, e che mi pare sia imprescindibile, è un rigoroso esame di accesso alla magistratura di legittimità, proprio per evitare

possibile tavolo di concertazione. Qualche giorno fa il senatore D'Onofrio, intervenendo immediatamente dopo il Ministro, diede un termine perentorio, dicendo: se entro martedì non ci dite cosa intendete fare, cesserà ogni possibilità di dialogo.

non solo perché porta il nome di un nostro Ministro, ma anche

prima di tutto dalla mia persona. Voglio lanciare proprio un messaggio alla maggioranza, poiché ritengo necessario un confronto su questa legge, così importante per il Paese. D'altronde, i riformisti dicono che siedono a sinistra

Si tratta di una riforma che incide sull'organizzazione interna della magistratura, tentando di ridisegnarne il sistema di accesso, in modo tale da recuperarne la professionalità, l'efficienza, l'indipendenza e l'imparzialità.

Sono stato il primo consigliere comunale della Lega, allora Lega Lombarda, e mi sono seduto in consiglio comunale a Varese nel 1985. Il nostro pensiero autonomista

fece scattare un avviso di garanzia nei miei confronti: dopo tre giorni mi trovai davanti ad un magistrato, che mi vietò espressamente

Nell'ambito del mio potere politico di consigliere comunale ritenevo di poter affermare quello che il mio movimento intendeva esprimere: tre giorni dopo, però, mi trovai davanti ad un magistrato. Ricordo ancora molto bene bene la situazione: vidi nella magistratura il braccio armato dello Stato, che voleva fermare all'inizio, sul nascere, un movimento che era l'espressione del mio popolo.

Penso che lo facciano molti senatori nati appena dopo la seconda guerra mondiale: l'intercalare il proprio dire con frasi in dialetto o in lingua locale è un qualcosa di naturale.

dei passi che ho subìto da parte della magistratura (perché poi di avvisi di garanzia il sottoscritto, per impegni politici, ne ha collezionati

al finanziere che stava stenografando il mio intervento. Ma il ragazzo, purtroppo per lui, era nato a Catania e non poteva dare nemmeno un aiuto al magistrato nella stesura del verbale.

quando il pretore di Saronno mandò 20 carabinieri presso il mio studio a sequestrare volantini e giornali (l'allora giornale «Lombardia Autonomista»).

pagarmi la campagna elettorale. Ancora adesso la questione non è stata chiarita e questa volta non sono mai stato chiamato dal magistrato, mai

politica, con un colpo di spugna cerca di fermare una riforma che ritengo indispensabile. Mi avvio a concludere il mio intervento e lancio un appello agli amici della sinistra: questa tecnica di Penelope, come io la chiamo, non porta da nessuna parte.

riscoperto, condiviso e portato a termine per il bene comune.

che vengono applicate in modo rapido, con criterio equo. Ma non solo questo: credo sia necessario anche che ogni utente della giustizia, ogni cittadino abbia la convinzione anche lui, come il contadino prussiano, di avere il suo giudice a Berlino. Non è facile avere una buona giustizia,

Ora, cosa è avvenuto negli ultimi anni del nostro Paese? Che invece di discutere di buone leggi, di applicazione rapida delle medesime, di equità ed imparzialità della giustizia, si è parlato soprattutto dei rapporti fra giustizia e politica, fra magistratura e Parlamento. Lo si è fatto in un modo un po' contrario alla storia, cioè difendendo non tanto la magistratura dall'invasione della politica, quanto il contrario, e lo si è fatto con una *vis* polemica sicuramente esagerata. Molto è venuto dagli anni di Tangentopoli: ricordiamo la enfatizzazione mediatica, il protagonismo di tanti magistrati che poi si sono trasferiti in politica e nelle Aule del Parlamento; ricordiamo soprattutto gli effetti di quei momenti: moltissimi indagati, processati attraverso i *media*, e poi tanti assolti; soprattutto ricordiamo la distruzione per via giudiziaria di partiti storici che, pur avendo enormi difetti, non meritavano quella fine. Ma ricordiamo anche fatti antecedenti e successivi: magistrati che, partecipando a feste di partito, tengono comizi, oppure che, commemorando la Resistenza, si spingono a paragoni sicuramente eccessivi fra i regimi di un tempo e il Governo di centro-destra di allora; ricordiamo magistrati che intervengono in via preventiva rispetto a leggi che il Parlamento si appresta a votare: immagino cosa succederebbe se io, in qualità di parlamentare, intervenissi nella mia città rispetto ad un processo in corso chiedendo questa o quell'altra sentenza; ricordiamo i documenti della magistratura, gli scioperi e via dicendo. Gli effetti di tutto ciò sono tanti: sono tanti: sicuramente un'invasione di campo da parte di una certa magistratura organizzata e militante nel settore politico; i dubbi, sempre più diffusi nei cittadini, sulla imparzialità dei magistrati; in ultimo, questa atmosfera e questo contesto, aggiunto ai ritardi storici e alla lentezza cronica della nostra magistratura, sia civile sia penale, provocano un calo di fiducia verso la magistratura nel suo insieme.

emanate molte leggi, ma non si è riusciti a fare quella riforma vera e profonda della giustizia sia civile, sia penale, con responsabilità che sono un po' di tutti: sicuramente della maggioranza, sicuramente dell'opposizione di allora, sicuramente del raccordo che c'era con una certa magistratura che pesava coi suoi giudizi e i suoi orientamenti su certe forze politiche. Ma qualcosa di buono è stato Questa riforma dell'ordinamento giudiziario, non fosse altro perché fa esistere qualcosa che doveva esistere già cinquant'anni fa

la separazione delle funzioni, che tende a produrre dei giudici più terzi e dunque più imparziali; il voler tendere ad avere dei magistrati più preparati, promossi per merito; la precisazione del ruolo delle procure e del Guardasigilli. Questo è stato realizzato, anche se non è stata una riforma sconvolgente.

Adesso, con la nuova legislatura, l'attuale maggioranza propone di bloccare tre decreti significativi di quella riforma e poi di operare delle consistenti modifiche.

Ma il blocco - come ribadito da tanti senatori dell'opposizione - significa una grossa interruzione della continuità istituzionale e denota troppo significativamente ed evidentemente come ci sia una volontà di apportare modifiche distruttive rispetto al testo approvato.

a discutere subito per migliorare, per sentire, per continuare questo discorso e questo confronto tra le forze politiche. Credo che il nostro atteggiamento sia corretto, sereno e costruttivo, in linea con quell'opposizione decisa ma responsabile che il nostro partito intende attuare su tutti gli argomenti importanti. Credo anche che sia il massimo che l'opposizione possa proporre. Invitiamo dunque la maggioranza a riflettere. Non vogliamo essere prevaricati da nessuno, siamo disponibili a collaborare - ripeto - e, se facciamo questa resistenza sulla legge dello scorso anno, la facciamo convinti

che serve con grande positività ed efficacia il Paese, che ha lasciato feriti e morti nel cammino della sua storia e che merita il nostro grande rispetto. Ripeto: opposizione e disponibilità.

la legge Castelli, questa riforma che porta il nome dell'ex ministro della giustizia, non ha prodotto effetti devastanti nonostante sia in vigore

Avrei potuto capire, e credo che anche i cittadini italiani lo avrebbero compreso, se questa riforma avesse realmente realizzato dei presupposti devastanti all'interno del sistema giudiziario,

Credo che l'intento sia un altro, perché non si può sospendere una legge che al suo interno, oltre alla delega per dieci decreti legislativi, contiene anche una norma che abroga totalmente il sistema di norme legislative precedenti in materia. Come ha ben detto il giorno che discutevamo della questione pregiudiziale il senatore D'Onofrio, non esiste in nessun caso la possibilità

che è sovrano e viene eletto per legiferare e quindi emanare leggi, si faccia invece dettare le regole da *lobby*,

dei cittadini e dobbiamo avere il coraggio di interpretare la nostra funzione nella correttezza massima; dobbiamo certamente ascoltare le associazioni, le categorie, ma soprattutto dobbiamo ascoltare i cittadini, dobbiamo guardare alle disfunzioni che le leggi che noi emaniamo creano all'utente finale, cioè al cittadino. Invece avviene che ci facciamo condizionare dalle *lobby*, come in questo caso: la sospensione che viene richiesta è un impegno elettorale, com'era stato un impegno elettorale il decreto Bersani in alcuni suoi contenuti, ad esempio nel caso delle farmacie, che dovevano essere date alle cooperative. In questo caso vi è stato un impegno per sospendere una legge che sicuramente, come per ammissione dello stesso senatore Castelli, non è la migliore delle riforme, ma certamente la prima riforma dopo

No, invece non è così: non c'è questa volontà. Vi è una volontà disfattista. Non è questo il primo caso. Anche in altre istituzioni, come le Regioni

coloro che vengono eletti sono interpreti delle esigenze dei cittadini, anche appartenenti a coalizioni diverse, quindi lavorano certamente per apportare dei miglioramenti. Anche in questo caso, io credo che una

Inoltre, signor Sottosegretario, non so che cosa ci proporrete successivamente, ma vorrei sapere una cosa. Parliamo, ad esempio, delle disfunzioni

strutturali: perché non si rivede il sistema organico e perché avviene che procure che hanno carichi di lavoro ridottissimi hanno in dotazione un personale quattro volte superiore alle procure che invece hanno un carico notevole? Perché non si provvede allo spostamento di risorse umane? Perché non si provvede a stanziare maggiori risorse laddove

nelle finanze dello Stato, però credo che il settore giudiziario non debba subire perdite finanziarie, perché non è possibile che i cittadini aspettino per avere giustizia venti,

Il sistema va cambiato e va cambiato notevolmente: noi dobbiamo avere il coraggio di farlo. Ci avete proposto questa sospensione per noi illogica; era più giusto, invece, iniziare a discutere immediatamente su quei decreti che bisognava correggere,

di intervenire nel condizionare le funzioni di altri organi: questo non è corretto. I magistrati sono funzionari dello Stato chiamati a far applicare le leggi che il Parlamento emana, non le leggi che loro vogliono che il Parlamento adotti! Non esiste che un magistrato possa intervenire sul dibattito in materia di separazione delle carriere: questa è una scelta che deve fare il Parlamento, non i magistrati!

però il Parlamento deve recuperare la propria dignità, quella dignità che gli appartiene e per la quale noi veniamo eletti. Dobbiamo avere il coraggio di assumerci le nostre responsabilità,

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, una norma chiarisce, meglio di altre, la cifra politica di questo scarno disegno di legge,

Qual è la norma la cui applicazione questa disposizione intende sospendere? È una norma contenuta non nell'ordinamento giudiziario riformato,

del Consiglio superiore della magistratura non può porre il magistrato togato uscente da queste funzioni in una posizione di privilegio ai fini delle funzioni che sarà chiamato a svolgere. Ora, l'articolo 3 del disegno di legge, sospendendo l'operatività di questa disposizione, riporta alla situazione *ante* 2002. Riporta, cioè, ad una situazione di fatto

prima domanda che rivolgo al Governo, se ha voglia di ascoltare e soprattutto di rispondere, è la seguente: che cosa c'entra questa norma con l'ordinamento giudiziario?

Ad essere maliziosi si potrebbe rispondere che la ragione sta nell'ennesima cambiale che il Governo nel suo insieme, ma il Ministro della giustizia in modo particolare, paga con questo provvedimento. Parlo di una cambiale perché per l'intera legislatura passata vi è stata una polemica continua sulle leggi definite *ad personam* salvo poi ammettere, a mezza voce, che più d'una di esse aveva un suo fondamento e una sua logica: penso per tutte alla riforma dei reati societari, conosciuta ingiustamente e falsamente come abolizione del falso in bilancio

consiglieri togati uscenti del CSM. L'intera politica con cui l'attuale Governo ha avviato la legislatura in materia di giustizia sembra caratterizzata dal pagamento di cambiali. È accaduto così verso l'area della criminalità con l'indulto, che sta causando effetti devastanti, basta chiedere al sindaco di Napoli: chiamo in causa un esponente politico che non sta accadendo, *mutatis mutandis*, con il presente disegno di legge di sospensione dell'ordinamento giudiziario. E la cambiale, come è accaduto per l'indulto, viene pagata danneggiando i diritti degli altri. gli altri sono i magistrati diversi dai sedici - lo ripeto, degnissimi - togati uscenti del CSM, che probabilmente hanno titoli e anzianità più qualificanti che però rischiano di essere - il rischio è più che concreto - sopravanzati nel momento dell'assegnazione delle funzioni. Il tutto con una formulazione normativa per la quale il senatore Calvi, anch'egli non appartenente ad Alleanza Nazionale, in sede di parere da parte della Commissione affari costituzionali ha scritto: «Si segnala l'opportunità di una diversa formulazione dell'articolo 3, tale da rispettare in forma più congrua la sequenza normativa, considerato che la norma abrogata è fatta rivivere senza intervenire sulla norma abrogante. L'intervento, infine, dovrebbe aderire in modo più appropriato alla natura generale e astratta del rapporto tra norma abrogata e norma attualmente vigente». La tecnica legislativa più elementare insegna che l'abrogazione di una norma in questo caso la sospensione del suo vigore - non ha un potere taumaturgico, cioè non può fare miracoli, non ottiene di per sé, come risultato, la resurrezione della norma antecedente. Non si può dire a una norma del 1990, modificata nel 2002: «Alzati e cammina, alzati e riprendi la tua efficacia». Volete perlomeno riscriverla? Non so se nei criteri di economicità che hanno caratterizzato la costituzione e la formazione di questo Governo rientri anche la micragnosità nella stesura delle norme. con la stessa tecnica legislativa, censurata da un esponente qualificato della maggioranza qual è il senatore Calvi in un momento qualificato (l'espressione del parere in 1ª Commissione permanente), si potrebbe dire: è sospesa l'applicazione delle norme del codice civile, rivivono le 12 Tavole, dal mio punto di vista, erano tutt'altro che spregevoli. È una norma incostituzionale. Sarà impugnata dagli interessati davanti al TAR e, attraverso questo, davanti alla Consulta, a fronte di ogni assegnazione di posti che veda concorrere consiglieri uscenti del CSM, qualunque sia l'esito del concorso. È incostituzionale perché non risponde a criteri di generalità e di astrattezza, visto che abbiamo 16 nomi e cognomi ogni 4 anni. Non risponde a criteri di eguaglianza per le ragioni che prima indicavo e non risponde al rispetto di quell'articolo 97 della nostra Carta fondamentale che richiama l'imparzialità dell'amministrazione. Non risponde a criteri di ragionevolezza perché se per un posto direttivo sarà preferito un magistrato meno anziano e meno virtualmente capace, ne ricaverà danno la razionalità del sistema. Non risponde - se mi si permette un fatto personale al criterio di eguaglianza, anche con riferimento agli altri magistrati che, in aspettativa in questo momento, si trovano a far parte di corpi elettivi.

a concorrere con criteri di minore preferenza rispetto al primo? Noi non vogliamo svolgere alcuna opposizione aprioristica e preconcetta. Diciamo soltanto: non vi piace l'ordinamento giudiziario che è stato approvato nella passata legislatura - ciò è legittimo cambiatelo, mostrateci un'ipotesi alternativa. Ricordo che nel 1996 l'allora Ministro della giustizia (era un signore che oggi è vice presidente della Consulta, il professor Flick)

e a questa paletta rossa nei confronti dell'ordinamento giudiziario. Perché un blocco secco? Perché - tutto ha una ragione - il Governo non ha avuto ancora tempo e modo di trattare compiutamente con l'Associazione nazionale magistrati su come riformare l'ordinamento giudiziario e ritengo che ce ne vorrà di tempo. E allora, non riuscendo ad arrivare ad un'ipotesi alternativa, è molto più comodo porre uno disinteressandosi - uso un eufemismo - delle conseguenze concrete che questo stop può avere nel quotidiano andamento della giustizia. Sarei veramente sorpreso se in questo ramo del Parlamento questa linea fosse condivisa da senatori che si sono sempre e motivatamente espressi nella direzione di rivendicare la piena libertà delle Camere a legiferare, anche in materia di giustizia, senza ricevere *input* da vertici di congregazioni togate. Sono ben consapevole che ogni riforma richiede la consultazione dei diretti interessati e deve puntare, nei limiti del possibile, a fare da eco alle loro esigenze, ma ciò è quello che i proponenti della riforma nella passata legislatura hanno provato a fare, perlomeno in una prima fase. anzitutto ripreso proposte relative all'ordinamento giudiziario che si inserivano in un filone che già era stato preso in considerazione all'epoca della Commissione bicamerale dalle varie bozze dette «Boato», dal nome del relatore all'interno della Commissione. Poi si è arrivati ad un momento, nel maggio del 2002, di possibile concreta convergenza con i vertici della magistratura associata per una riforma adeguata anche alle loro esigenze. Per questioni assolutamente interne a quell'associazione, un accordo quasi raggiunto fu mandato all'aria; si arrivò ad uno sciopero, il primo di una serie, che inaugurò una sequela di proteste dall'esibizione della Costituzione ai girotondi e così via. Questo per dire che vi è stata l'occasione per giungere ad una riforma della giustizia parzialmente diversa da quella approvata in via definitiva, certamente più vicina alle esigenze del mondo della magistratura, ma questa occasione è stata respinta dagli stessi interessati.

giudiziario, l'allora segretario dell'Associazione nazionale magistrati paragonò il Governo di centro-destra al regime di Mussolini. Tale affermazione fu pronunziata non in un bar, ma nella sede del congresso dell'Associazione nazionale magistrati ed ebbe echi anche in Parlamento. mi chiedo se sia proprio così. Si può anche non condividere nessun aspetto di questa riforma, ma si può avere il gusto e la soddisfazione di discuterla nel merito? Si è protestato, per esempio, perché la riforma vieta ai pubblici ministeri di diventare giudici nello stesso distretto. Gradirei sapere quale pericolo per le libertà democratiche del Paese derivi da questa previsione.

Non solo l'odiato centro-destra, ma gran parte della cultura italiana ritiene che una moderata articolazione di carriera basata su concorsi stimolerebbe la professionalità e la formazione professionale dei giudici e valorizzerebbe la Corte di cassazione. Ma anche su questo versante si sostiene che sottoporre i giudici alla valutazione di una Commissione tecnica, benché espressione del CSM, equivale a riesumare Salazar e Pinochet. E ancora, è golpistico fare chiarezza sugli illeciti disciplinari e sulla procedura per sanzionarli?

poi un profilo sul quale dovremmo intenderci in Parlamento e riguarda la pretesa, non dichiarata ma reale, che la gestione politica del nostro Paese avvenga nelle aule di giustizia; la pretesa, cioè, di considerare che il compito dei magistrati non è il controllo sui singoli atti illeciti commessi dai politici - il che è doveroso - ma è il controllo della politica nel suo insieme.

sulla base del tempo e dello spazio. La custodia cautelare non è intesa alla stessa maniera a Milano, a Roma o a Bari. In alcuni processi viene utilizzata la presunzione del «non poteva non sapere», e in altri ciò delle medesime carte alcuni giudici assolvono e altri condannano. Ora quest'alternanza fa onore all'indipendenza della magistratura, ma da essa non possono dipendere i destini politici del Paese. Gli italiani leggono i giornali, guardano la televisione e constatano che magistrati eminenti, spesso responsabili di processi delicati e difficili,

si può condividere o no la riforma Castelli, si può discutere, entrare nel merito - ed auspichiamo che ciò avvenga - ma dovrebbe essere un dato di comune condivisione che il magistrato deve essere ed apparire imparziale, che deve avere una professionalità seria e verificata, che non può comportarsi come un politico di professione. Con questo blocco il Governo, e la maggioranza che lo sostiene, non aiuta la magistratura, anzi concorre con fatti concludenti a confermare che il rischio più forte per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura proviene dall'interno della stessa magistratura.

l'applicazione delle leggi, non nella sostanza i diritti, non procurando dei vantaggi ad alcuni cittadini a scapito di altri, ma cercando di normare e di mettere ordine nella macchina dell'amministrazione e di definire anche come si dovrebbero svolgere le carriere. Velocemente vorrei ripercorrere, in sintesi, i grandi titoli di questo stravolgimento della giustizia, come è stato presentato da questo Governo e dai *mass* *media*, evidentemente molto vicini ad esso. Come la separazione delle funzioni prima di questo decreto? L'aspirante magistrato, dopo un anno di tirocinio da uditore, partecipava al concorso per entrare in magistratura e chiedeva di fare il giudice o il pubblico ministero. Molti, soprattutto in primo grado, facendo domanda al CSM, cambiavano funzione anche più volte. Con questo decreto si prevede che nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante magistrato deve scegliere tra giudice o pubblico ministero. Il concorso prevede anche un colloquio di idoneità psico-attitudinale che può indirizzarlo verso una funzione o l'altra. La sua scelta definitiva avviene dopo cinque anni. Per cambiare funzione deve sostenere un esame orale e frequentare un corso di formazione presso la Scuola della magistratura ottenendone una valutazione positiva. Inoltre, dovrà cambiare distretto giudiziario e qui forse sta lo scandalo. Come era si occupava della formazione delle toghe organizzando dei corsi non obbligatori. Non esisteva una scuola per la magistratura come è oggi. La formazione per gli uditori, ma anche per l'aggiornamento professionale e la valutazione dei magistrati è compito della Scuola superiore per la magistratura e i corsi sono obbligatori ogni cinque anni. Al termine del corso viene formulata una valutazione. Il comitato direttivo è composto dal primo presidente e dal procuratore generale della Cassazione, da due magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno 15 anni di servizio nella professione, da un professore universitario e da un membro nominato dal Ministro della giustizia. Soltanto

di poter esprimere la sua opinione sulle capacità di un magistrato, non sul modo di amministrare la giustizia? Come era la carriera? L'avanzamento di carriera avveniva automaticamente, per anzianità. In pratica, dopo 13 anni si accedeva alla Corte d'appello e dopo 28 alla Cassazione senza concorsi. Anche senza svolgere effettivamente quelle funzioni, lo stipendio veniva adeguato. Com'è Chi vuole può continuare a seguire la vecchia strada, un numero limitato di posti (30 per cento) è a disposizione di coloro che vorranno accelerare la propria carriera, sostenendo un concorso che prevede la risoluzione (scritta) e la discussione (orale) di uno o più casi pratici che riguardano il proprio lavoro di magistrato. magistrato. Come era l'organizzazione delle procure? II capo della procura dava delle direttive e organizzava il lavoro dei suoi aggiunti e sostituti, ognuno dei quali era titolare dell'azione penale, aveva una sua autonomia nelle inchieste e poteva rilasciare dichiarazioni alla stampa. Solo in alcuni casi poteva avocare a sé un'inchiesta. Come è con il decreto da bloccare? Il capo della procura ha più poteri. E' l'unico titolare dell'azione penale che "delegherà" agli altri pubblici ministeri. Una delega revocabile per l'assegnazione dei procedimenti, in caso di divergenza o inosservanza dei criteri indicati, con una comunicazione alla Cassazione. E' l'unico a tenere i rapporti con i *mass media.* Questo è uno scandalo perché tutti oggi vogliono parlare con le televisioni. Come era l'azione disciplinare? L'azione disciplinare era facoltativa e ne erano titolari il procuratore generale della Cassazione e il Ministro della giustizia. Veniva applicato il codice del 1930 e non esisteva una tipizzazione dei reati. Come In caso di illeciti disciplinari l'azione del procuratore generale della Cassazione diventa obbligatoria e non più facoltativa. Il Ministro della giustizia può opporsi al non luogo a procedere solo per i casi da lui stesso promossi. Quindi, non ha un potere assoluto.

II Consiglio superiore della magistratura autorizzava gli incarichi extragiudiziari per i magistrati, senza alcun obbligo di pubblicità. Come è oggi? Gli incarichi extragiudiziari alle toghe, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura, devono essere pubblicizzati in un elenco ogni sei mesi. I magistrati, inoltre, non possono iscriversi a partiti politici né partecipare ad attività che li possano condizionare o appannarne l'immagine. Sinceramente trovo che lottare contro una regolamentazione interna all'organizzazione - che nulla a che vedere con l'applicazione della legge - per migliorarla ed avvicinare di più la classe della magistratura alla normalità degli esseri umani che abitano in questa Nazione non solo non sia disdicevole ma sia doveroso. Trovo meno doveroso, invece, leggere alcune applicazioni di una recente sentenza del 18 settembre 2006 della Corte suprema di Cassazione, prima sezione penale, nella quale si vede invece quale sia il pensiero della magistratura. Con quella sentenza il tribunale di Roma ha assolto, perché il fatto non sussiste,

trovata nel territorio dello Stato, da cui era stata espulsa mediante ordine di allontanamento. Il giudicante ha fondato la decisione su una duplice argomentazione. Doveva ritenersi sussistente il giustificato motivo che esclude la punibilità del fatto (essere clandestini con un'ingiunzione di allontanamento dal territorio nazionale), avendo l'imputata dichiarato di essere sprovvista del denaro occorrente al rimpatrio. Circostanza plausibile - sentite perché - essendo emerso che alloggiava presso uno scalo ferroviario ed essendo risultato che non aveva compreso appieno il contenuto del provvedimento esecutivo dell'espulsione, tradotto soltanto in inglese, in quanto durante il dibattimento aveva dovuto essere assistita da un interprete di lingua romena. Nella nostra Repubblica, patria del diritto, basta dimostrare di non avere mezzi di sussistenza e di non comprendere la lingua italiana per essere scagionati da qualunque reato. Credo che ciò gridi allo scandalo, e non normare l'organizzazione interna che porta alle cariche supreme della magistratura, che nulla ha a che vedere con l'intromissione da parte del Governo e dei due rami del Parlamento nell'amministrazione della giustizia. Mi piacerà vedere, insieme a tutti i nostri colleghi che hanno volentieri e plaudendo approvato il decreto Castelli, quali saranno le esilaranti e fantasmagoriche modifiche che la parte più politicizzata della magistratura vi apporterà, dopo averlo congelato e lasciato marcire in un *freezer*, togliendo anche la spina, cosa accadrà all'organizzazione della magistratura. Prepariamoci, perché probabilmente, seduti al tavolo dove ora siede lei, Presidente, ci sarà un rappresentante della magistratura nei prossimi Parlamenti. *(Applausi dei

*(DC-PRI-IND-MPA)*. Signor Presidente, senatori, signor rappresentante del Governo, mi sia consentito iniziare con la citazione di un documento di qualche giorno fa, che molto attiene alla nostra discussione. Quel documento - il cui autore

rinnova la sua richiesta al Governo e al Parlamento di fronteggiare, con i mezzi istituzionali di cui dispongono, la vera e propria emergenza determinata, nell'ordinamento giudiziario e nel funzionamento della giurisdizione, dall'entrata in vigore di una legge di riforma che continua a giudicare sbagliata, paralizzante e controproducente; ribadisce di non essere in alcun modo a favore di sospensioni ripetute o illimitate e di volere in tempi brevi l'approvazione di una riforma dell'ordinamento giudiziario ragionevole e coerente con i princìpi costituzionali; sottolinea l'assoluta necessità che il previsto intervento normativo sia adottato prima del 28 ottobre 2006, al fine di scongiurare la separazione di fatto delle carriere giudicante e requirente che a quella data rischia di verificarsi e l'avvio di un sistema di organizzazione della carriera dei magistrati contrario ai princìpi costituzionali ed alle esigenze di efficacia e funzionamento della giustizia». Infine, il Comitato centrale «dà mandato alla Giunta

un Comitato centrale, una Giunta che dà esecuzione, alcuni punti di premessa e un dispositivo finale; a firmare tale documento è l'Associazione nazionale magistrati, il cui Comitato centrale si è riunito sabato scorso.

il Parlamento nella scorsa legislatura ha approvato una riforma ed oggi un partito extraparlamentare, che non ha consenso nel Paese e non può candidarsi alle elezioni,

«Avvenire» del 6 settembre, Giuseppe Gennaro, presidente della suddetta Associazione nazionale magistrati (cioè di quel partito extraparlamentare che influisce e determina le volontà del Parlamento, essendo costituito, in quanto partito extraparlamentare, fuori dalle regole della nostra Costituzione), dice: «La riforma dell'ordinamento giudiziario va sospesa: se non ci sarà uno sviluppo alla ripresa dei lavori parlamentari, non resteremo a guardare». Sarebbe stato interessante sapere dal presidente Gennaro che cosa intende con «non resteremo a guardare». Colleghi, provo a sollecitare in voi una riflessione. Se a pronunciare parole di questo genere fosse il più alto rappresentante sindacale della Polizia di Stato o il più alto rappresentante del COCER dei Carabinieri o un qualche generale dell'Esercito o di qualunque altra Arma, vi sarebbe una reazione della politica e dell'opinione pubblica che chiamerebbe questi atti insurrezione, *golpe*, attentato alle prerogative parlamentari. Invece, il fatto che lo facciano il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati e l'Associazione nazionale magistrati stessa, con quel tono tipico dei partiti politici, passa come un fatto di normalità e anzi si fa di tutto per rispondere a questo *diktat*. Signor Presidente, questa è la situazione in cui ci troviamo. Il Ministro - che purtroppo non è presente oggi - aveva cercato in qualche misura di temperare tale quadro, intanto facendo presente che la maggioranza in Senato su questo provvedimento aveva qualche difficoltà ulteriore rispetto alle innumerevoli difficoltà che ha su tutti gli altri. Ma di tutta risposta il segretario dell'ANM, il giorno 7 settembre (lo ha pubblicato «Il Sole 24 Ore») ha detto: «Il dialogo con l'opposizione non può diventare un alibi per giustificare l'inerzia del Governo e della sua maggioranza».

e potrebbe richiedere alle forze della sua maggioranza una coerenza. È vero, infatti, che nel programma dell'Unione c'era scritto: «È necessario rimuovere tutti gli aspetti del nuovo ordinamento in stridente contrasto con i princìpi costituzionali, anche adottando provvedimenti di sospensione». L'ha ricordato di recente un magistrato, il dottor Giancarlo Caselli (di cui si ricordano più le gesta politiche e meno

Vorrei solo far notare che lo scorso Parlamento aveva sottoposto la riforma al vaglio di costituzionalità, approvandola in tutte le fasi in cui il nostro Regolamento e il Regolamento della Camera impongono un esame della costituzionalità delle norme che vanno a discutersi e ad approvarsi. Ma c'è di più. Il 16 dicembre 2004, con messaggio motivato, il Presidente della Repubblica rinviava questa riforma alle Camere, sottoponendo al Parlamento una serie di punti che a suo avviso erano in contrasto - non stridente, diceva il Presidente, ma in contrasto - con la Carta costituzionale. Ebbene, il Parlamento ha recepito quel messaggio del Capo dello Stato, ha modificato le norme su cui il Capo dello Stato aveva chiesto di intervenire e, a quel punto, ha varato un nuovo provvedimento, diverso da quello in prima lettura, che il Capo dello Stato ha promulgato, sancendo in questo modo che la nuova versione era assolutamente aderente ai princìpi costituzionali, perché altrimenti, trattandosi di un nuovo testo, non era impedito nella Facoltà di rispedirlo ulteriormente al mittente qualora il nuovo testo non avesse soddisfatto le indicazioni giunte nel messaggio motivato.

che conclude, un po' sibillino nei confronti del Governo e della maggioranza parlamentare, dicendo che se la riforma Castelli non verrà sospesa e poi smantellata - ed è importante la citazione - «c'è il rischio - magari inconsapevole - di ritrovarsi in un'altra compagnia (quella di Licio Gelli) e potrebbe suonare - paradossalmente - un po' come darla vinta al "venerabile" piduista». Dunque abbiamo così preavvisato il ministro Mastella e tutti coloro che nella maggioranza hanno qualche perplessità, che di lì a poco, se non ottempereranno a questi *diktat*, saranno tacciati di essere - come dire? - piduisti di ritorno? Piduisti di seconda fila? Piduisti inconsapevoli? Comunque piduisti. Saranno cioè demonizzati come coloro che coloro che vogliono sovvertire l'ordine costituzionale, mentre ci troviamo di fatto in una sovversione dell'ordine costituzionale da parte dell'ordine giudiziario e della sua espressione associata, che si chiama Associazione nazionale magistrati, con i suoi documenti ufficiali che bisognerebbe sottoporre a qualche autorità, se esistesse una autorità indipendente in questo Paese in tale ambito. Ma non basterebbe il tempo che abbiamo a disposizione in questo dibattito, signor Presidente, colleghi, per analizzare quello che è il perverso intreccio che c'è stato tra parte della magistratura e parte della politica, la sinistra segnatamente, ed è quello che provoca questa soggezione che il Governo vuole imporre al Parlamento nei confronti della magistratura. Meglio di me potrebbero spiegarlo due colleghi che fanno parte di quest'Aula, che purtroppo non vedo, che sono i senatori Andreotti e Mannino, i quali hanno subito e sono stati vittima di quel perverso intreccio tra parte della magistratura e parte della politica. Il Ministro ha cercato in qualche misura di non rimanere ostaggio, di non restare stritolato in questa morsa e ha tentato di dare un colpo al cerchio ed uno alla botte in questi mesi. Ad esempio, il 7 agosto ha disposto, per accontentare l'Associazione nazionale magistrati che lo chiedeva da tempo, che la citazione dell'articolo 101 della Costituzione («La giustizia è amministrata in nome del popolo») fosse rimossa dalle aule di giustizia. giustizia. Abbiamo avuto cioè una contestazione da parte della magistratura perché una frase, che apre un articolo della Costituzione, era stata posta come massima cui attenersi nelle aule della giustizia italiana.

che è arrivata fino a voler cancellare una massima di norma costituzionale dalle Aule di giustizia? Ed è assolutamente scandaloso che in questo il Ministro si sia assoggettato, tentando forse di placare l'animo, che ovviamente non è stato placato, di una magistratura che cerca una rivalsa politica contro le riforme e contro una parte politica che quelle riforme aveva proposto al corpo elettorale, aveva avuto un mandato per realizzarle e le aveva realizzate. Ma per dare un colpo alla botte, il Ministro ha, ad esempio, nominato a presiedere la Commissione per la riforma del codice penale l'avvocato Giuliano Pisapia, già membro del Parlamento, esponente del Partito di Rifondazione Comunista, che, peraltro, prima delle elezioni del 9 e 10 aprile, era stato candidato a Ministro della giustizia dell'eventuale futuro Governo dell'Unione. L'avvocato e onorevole Pisapia, a proposito della riforma dell'ordinamento giudiziario, aveva pronunziato una frase che voglio riportare in questo dibattito e che mi sento totalmente di sottoscrivere. Egli ha affermato: «La Casa delle Libertà aveva proposto la separazione delle carriere nel suo programma elettorale nel 2001 e poi non l'ha realizzata nella sua riforma». E' vero: è stata una mancanza, abbiamo fatto meno di quanto ci eravamo impegnati a fare con gli elettori. «Nel programma presentato dal centro-sinistra» - continua Pisapia - «proponiamo una più netta separazione delle funzioni in modo da evitare che possa svolgere la funzione di giudice chi qualche mese prima aveva fatto il Pm nello stesso tribunale e nella stessa aula di giustizia».

dopo qualche intervista giornalistica di carattere generale ha dovuto fare marcia indietro. Egli ha dovuto dire che per il Governo devono essere cambiate le norme sull'organizzazione delle procure, sulle carriere, sulla formazione professionale e sui procedimenti disciplinari.

Eppure da parte nostra non era giunta una preclusione a un proficuo rapporto con la maggioranza e il Governo anche, eventualmente, per correggere la riforma. Ricordo la nostra proposta

il Parlamento, i rappresentanti della sovranità popolare avranno piegato la loro testa sotto i colpi prepotenti, e aggiungo, *extra legem* della casta dei magistrati costituitasi ancora una volta in un partito fuori dalle regole e contro la Costituzione.

prendere la parola in un dibattito così importante è sempre un momento di grande rilievo, che contribuisce a mio parere a formare, anche a livello parlamentare, quel senso comune di idee, di progetti e di obiettivi da raggiungere. Ho ascoltato con grande attenzione l'intervento del ministro Mastella.

una legge che deve entrare in vigore da subito per garantire la funzionalità di un servizio importante per il nostro Paese? In più occasioni abbiamo avuto modo

di revisione. Invece, il ministro Mastella credo non abbia avuto la possibilità di dare questo tipo di garanzie sui punti che abbiamo posto.

che mettesse al centro della discussione politica la diversità e l'autonomia dei poteri dello Stato. Ho ascoltato dai colleghi che probabilmente su questi temi occorrerà proporre un dibattito culturale per valutare se l'attività del legislatore nel nostro Paese su queste materie, sulla giustizia in particolare, debba

per garantire al nostro Paese quel livello di legalità di cui credo abbia bisogno. Davanti a queste nostre osservazioni ci siamo trovati di fronte ad una disponibilità a parole, nei fatti non abbiamo però riscontrato da parte del Ministro, del Governo e anche della maggioranza la disponibilità a discutere e ad entrare nel vivo

(una gestione quotidiana che a mio parere non porta da nessuna parte), con una politica di ampio respiro, sul risanamento economico, sulle riforme, sulla legge elettorale, legge elettorale, cioè sulla revisione delle regole e sulla ristrutturazione della politica in generale, potremmo trovare delle perché gli interessi non sono di una maggioranza o di una opposizione ma sono del Paese. Il nostro senso di difesa delle istituzioni, di responsabilità politica - in politica estera lo abbiamo dimostrato in più occasioni - la nostra coerenza sono la garanzia che la nostra volontà non è quella di incidere sulla sopravvivenza più o meno lunga di questa maggioranza, ma di affermare, ancora una volta qualora ce ne fosse bisogno, che davanti agli interessi generali del Paese, la nostra disponibilità è autentica. Davanti a questo noi ci ritroviamo prigionieri in un bipolarismo in un bipolarismo che da politico è diventato per blocchi elettorali, dove le esigenze delle estreme, delle corporazioni, degli interessi di parte, prevalgono prevalgono sull'interesse generale. Ecco, senatore Brutti e amici del Governo, io credo che questa sia stata un'occasione mancata.

che questo sia il contesto per entrare negli aspetti più tecnici, che si parli e si richieda un voto che non ritengo opportuno in questo momento storico. Il collega Castelli, tra l'altro,

può confrontare. Noi abbiamo posto il problema della separazione delle carriere: si tratta di problemi che vanno affrontati non a colpi di maggioranza ma convergendo con una comune volontà, anche da parte dei magistrati, per migliorare il servizio nel nostro Paese. non possiamo consentire che ci siano invasioni di campo, signor Presidente. Invasione di campo significa che, quando il Parlamento discute, non ci possono essere interferenze così forti.

Attendiamo anche le dichiarazioni del Governo e ci riserviamo, ovviamente, di fare ulteriori valutazioni, se da parte del Governo stesso ci saranno indicazioni di disponibilità

il disegno di legge che stiamo esaminando ha come obiettivo principale, nel sospendere la riforma dell'ordinamento giudiziario approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, dopo un lungo *iter*

introduce la separazione delle funzioni dei magistrati. Noi peraltro avremmo voluto la separazione delle carriere, questo era

dovremmo andare verso la separazione delle carriere. Siamo almeno riusciti ad approvare la separazione delle funzioni dei magistrati in modo da impedire un'eccessiva contiguità tra coloro che sostengono l'accusa

contiguità tale per cui c'è spesso da dubitare che il giudice si senta veramente terzo e veramente

espressione della volontà popolare, gradirebbero di godere di una loro indipendenza. Purtroppo, di fronte ai *diktat* che vengono dall'Associazione nazionale magistrati, o da altre associazioni di magistrati o da singoli magistrati, che però per il loro nome e, soprattutto, per il loro potere reale hanno di per sé una certa forza, mi pare che il

Qualche giorno fa c'è stata una sentenza della Cassazione nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi nella quale si è

certe associazioni di magistrati particolarmente attive nell'interessarsi al nostro lavoro di legislatori - e non so quanto attive nell'interessarsi al loro ruolo di magistrati,

Va ricordato che l'ordine giudiziario non esprime in nessun modo la sovranità popolare, poiché nella magistratura si entra per concorso mentre in Parlamento si entra per elezione, per scelta del popolo, al quale al quale in base al primo articolo della Costituzione, appartiene la sovranità. È curiosa questa gelosia della separazione, che è una gelosia a senso unico.

abbastanza politica. In essi si parla, in particolare, della protezione dei diritti degli immigrati e dei meno abbienti in una prospettiva di emancipazione sociale dei più deboli, del sostegno all'integrazione comunitaria ed europea - che non sapevo fosse una prerogativa dei magistrati

l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, sancita nel primo comma dell'articolo 104 della Costituzione. Ciò che viene sempre dimenticato è l'articolo 101 che, guarda caso, è il primo articolo che riguarda la magistratura, e riporta che «La giustizia è amministrata in nome del popolo» (del quale, peraltro, bisognerebbe ricordarsi qualche volta), mentre al secondo comma recita che «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Allora la legge dovrebbe essere applicata.

abbiamo assistito troppo spesso ad un uso della legge che viene applicata e disapplicata a seconda di ragionamenti politici. Io allora mi chiedo: se è reato definire politica una sentenza, non dovrebbe anche essere un reato definire contraria alla giustizia una legge? Non dovrebbe anche e soprattutto essere reato non applicare questa legge, magari farlo dichiaratamente, come a volte si trova in certi documenti fatti circolare da associazioni dei magistrati? Lo stesso sito di Magistratura democratica riporta antichi documenti di questa associazione, nata nel lontano 1964,

l'Assemblea nazionale di Magistratura democratica approvò una mozione che aveva delle frasi che sono forse un tantino politiche. Ad esempio questa: «...per la determinazione della linea politica della corrente vi è la convergenza su alcune acquisizioni fondamentali che si identificano nel riconoscimento: a) della caratteristica di classe della giustizia» - allora scopriamo che la giustizia è di classe per un'associazione di magistrati - «b) delle possibilità di fornire un contributo reale all'avanzamento del movimento popolare» (qui bisogna fare un po' di filologia nel 1971 per movimento popolare si intendeva sostanzialmente l'insieme della sinistra, che andava dal PCI fino alle frange collocate ancora più a sinistra le quali hanno anche intrapreso attività non più politiche, ma di altro tipo) «anche attraverso una nuova politica della giustizia» e, sempre in questa mozione approvata da Magistratura democratica, «c) che i problemi giudiziari non devono essere ridotti a meri problemi tecnici..., ma devono essere portati all'interno di tutto il movimento» (il "movimento popolare" del punto b) per «avviare un processo di riappropriazione popolare dei temi della giustizia». anche che bisogna rendere «funzionale alle esigenze di eguaglianza, partecipazione sociale, economica e politica delle classi lavoratrici» la «teoria e la prassi giudiziaria(...) attraverso la utilizzazione di tutte le contraddizioni del sistema democratico, non per mediarlo» (il sistema democratico, è scritto) «al fine di una razionalizzazione del sistema, ma per valorizzare gli elementi che possono portare al superamento del sistema stesso». Questo non è il proclama di qualche folle, di qualche singolo, ma è una mozione approvata da un'associazione che mi pare ha oggi il 25 per cento nelle elezioni per gli organi della magistratura e che all'epoca credo avesse un sostegno, forse un po' inferiore, ma comunque importante.

dichiarò che «per l'attuazione delle linee politiche» (sono loro a dirlo) «l'azione» (sempre della magistratura) «deve svolgersi sia all'interno che all'esterno dell'ordine giudiziario attraverso(...) la ricerca di collegamenti con tutte le forze politiche, tradizionali e non, della sinistra». tradizionali, ci si riferisce al Partito comunista e ad altri antichi partiti, mentre le forze non tradizionali in quegli anni stavano per accingersi ad attività di cui poi la magistratura ha dovuto interessarsi perché erano un tantino al di fuori della legge. Il 4 aprile 1973 l'Assemblea nazionale di Magistratura democratica approvò una risoluzione in indicava la necessità di costruire «un rapporto costante e articolato con le forze politiche e sindacali della sinistra(...) che consenta di ricercare(...) obiettivi politici(...) in un quadro strategico unitario inteso a battere il disegno reazionario e di ristrutturazione neocapitalista». Devo dire che questo vecchio armamentario vetero-marxista credevo fosse scomparso negli anni Settanta, mentre con questa legislatura ho imparato che ancora c'è, sentendolo a volte riecheggiare

sosteneva la necessità di «un impegno globale di Magistratura democratica per un crescente allargamento dei consensi all'interno e all'esterno della magistratura sulle linee sopra indicate» Nello stesso numero del giornale "Magistratura democratica", che riportava doverosamente questo documento ufficiale dell'Associazione, è un articolo di Pierluigi Onorato, un magistrato che ha scritto moltissime sentenze nella sua carriera, alcune delle quali riguardanti persone che oggi sono nostri colleghi Onorato sosteneva «l'esigenza sempre più avvertita all'interno e all'esterno del mondo giudiziario» che «questa frangia di magistrati democratici superi la fase della testimonianza per innescare un processo politico che investa tutta l'istituzione e assuma un valore per tutto il movimento», ossia il movimento prima menzionato, che era sostanzialmente l'insieme della sinistra. «Il momento presente impone a tutti una crescita politica, cioè il superamento dello spontaneismo». Basta quindi andare ciascuno per conto proprio, magari facendo sentenza in nome della legge. riferimento inoltre alla «continua preoccupazione delle implicazioni strategiche dei propri comportamenti: in una parola un approccio politico».

che porterebbe ai quadri democratici della magistratura a recuperare e difendere i valori della professionalità senza uno stretto legame col movimento. Occorre cementare nessi profondi tra movimento democratico» - cioè la sinistra - «e magistratura. È necessario approfondire rigorosamente i contenuti dell'azione politica perché siano sempre sorretti da una lucida consapevolezza strategica e verificati sulla base di questa». egli propone delle «mosse per far avanzare il fronte di lotta delle classi lavoratrici verso trincee finora riservate al nemico di classe». Alla luce di che possa limitare la possibilità di alcuni magistrati di fare politica con le loro sentenze - e spero che quanto rimane dell'articolo 68 della Costituzione sia sufficiente a proteggere ciò che sto dicendo da azioni di magistrati - se si può fare qualcosa per limitare quest'uso, che considero spudorato ed esplicito, della della magistratura per fare politica, credo che dovremmo davvero fare di tutto perché ciò avvenga. Nella scorsa legislatura l'abbiamo fatto; avremmo voluto fare di più, ma la riforma che oggi si vuole sospendere faceva grandi passi in questa direzione. come si faccia ad affrontare serenamente un processo se si sa che un magistrato, giudice o inquirente

Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, una premessa innanzitutto perché c'è da rimanere veramente allibiti ogni qual volta l'uno o l'altro esponente dell'opposizione interviene in Aula mettendo fortemente in discussione il ruolo e le decisioni dei senatori a vita. Poiché anche la settimana scorsa si sono ripetutamente verificati interventi di tal genere anche in occasione del voto sulla sospensione dei decreti in materia di ordinamento giudiziario, ritengo di dover dire due parole pur convinto che i senatori a vita non abbiano certo bisogno di difesa d'ufficio. Peraltro, soltanto due parole perché la semplice lettura della Sezione I del Titolo I della Parte II della nostra Costituzione fuga qualsiasi dubbio. I senatori a vita fanno parte a pieno titolo del Senato. In quanto membri del Parlamento rappresentano anch'essi la Nazione - articolo 67 - ed esercitano la loro funzione senza vincoli di mandato. Questo dice la nostra Costituzione, questa è la nostra Costituzione! Se non si è d'accordo esistono mezzi, strumenti e vie per modificarla. Che vengano presentati nuovi disegni di legge in materia e se ne discuterà, ma fino ad allora, fino all'approvazione e all'entrata in vigore di nuove norme, sarebbe il caso di smetterla con polemiche inutili, sterili, che vogliono essere soltanto propagandistiche o al limite dell'intimidazione, di smetterla di dire, come fa il senatore Schifani, sbagliando in diritto e in fatto, che l'allora Presidente della Repubblica, oggi senatore a vita, letteralmente votò quel testo e oggi si troverebbe, chissà per quale motivo poi, in situazione di conflitto. Vengo ora all'oggetto specifico del disegno di legge n. 635. Sono d'accordo con il senatore e presidente Francesco Cossiga quando dice che bisogna distinguere tra Associazione nazionale magistrati e magistratura. Ha ragione. Commentavo questa affermazione già in sede di Commissione giustizia. Sono due entità distinte, ma a noi sta a cuore non l'Associazione nazionale magistrati, ma la magistratura come organo costituzionale, sta a cuore l'efficienza e l'efficacia dell'attività giudiziaria. Èper questo motivo che, per tutelare la magistratura e quindi noi stessi in quanto cittadini - tutti i cittadini - bisogna impedire che mantengano la loro efficacia questi tre decreti legislativi, causa di confusione, di caos, di rischi di blocco dell'attività di organi costituzionali come il CSM, come denunciato pubblicamente dall'attuale vice presidente del Consiglio superiore della magistratura. Viene posta di sovente anche in quest'Aula una domanda. Ma è utile sospendere tutto? In questa situazione giuridica di fatto la risposta non può che essere positiva per due ordini di motivi. primo luogo, perché si possono determinare situazioni immodificabili, irreversibili, in materia di concorsi, di carriera, di azioni disciplinari, di interventi autoritari dei capi delle procure, in materia di separazione di funzioni secondo luogo, perché è in corso di presentazione un nuovo testo, sia da parte del Ministro della giustizia, come annunciato in Aula, sia da parte del Gruppo L'Ulivo, come segnalato più volte anche in sede di Commissione giustizia. Per quanto concerne ancorail primo ordine di motivi, va risposto che plurimi sono gli effetti - sarebbe da aggiungere ovviamente - già prodotti dai tre decreti per i quali si chiede la sospensione, innanzitutto con riferimento al primo dei tre da sospendere, il decreto legislativo n. 106, relativo alla rigida gerarchizzazione degli uffici del pubblico ministero. Varibadito che sono entrate in vigore norme che si pongono decisamente in contrasto con la nostra Carta costituzionale. Il primo e principale *vulnus* alla nostra Costituzione è generato proprio dalla dizione letterale dell'articolo 1, lì dove il procuratore della Repubblica viene definito letteralmente titolare esclusivo dell'azione penale.

e ogni sostituto procuratore è un pubblico ministero, un magistrato autonomo e indipendente, il quale dunque autonomamente deve avere la titolarità dell'azione penale. L'articolo 104 poi definisce la magistratura un ordine autonomo e indipendente e quindi ogni magistrato è autonomo ed indipendente. Il *vulnus* costituzionale introdotto sulla questione dalla controriforma Castelli già produce i suoi effetti ogni giorno, in ogni procura della Repubblica in materia di assegnazione di fascicoli, di gestione delle indagini e della polizia giudiziaria. legislativo n. 106 si scontra con un'altra norma di rango costituzionale, l'articolo 109, che dispone che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Quindi, ogni singolo magistrato di una procura può disporre dell'autorità giudiziaria. Ma se il titolare esclusivo dell'azione penale è il procuratore della Repubblica, allora ricordo come non io peraltro, ma un senatore esponente della Lega, il senatore Davico, in Aula la settimana scorsa, abbia parlato letteralmente di capi ufficio non all'altezza del compito. E in questi casi, per qualsiasi motivo si possano verificare (di età, di salute, di incapacità o anche indolenza), è evidente il danno gravissimo che si può arrecare ad indagini complesse e delicate come, peraltro, già in sede di Commissione di giustizia ricordavo, citando fatti concreti e specifici, e come benissimo ha ricordato in Aula il senatore D'Ambrosio. Non dimentichiamo poi un aspetto fondamentale dell'intera questione: il nostro sistema giudiziario è un modello di potere diffuso; modello che appare il più idoneo per una democrazia moderna come la nostra, che prevede delicati meccanismi nell'equilibrio tra i vari poteri dello Stato ed anche all'interno di questi stessi poteri. agli altri due decreti che vogliamo sospendere, nn. 109 e 160, sono ancora più evidenti i danni gravi ed irreparabili che si possono verificare proprio perché si parla di un decreto in materia di concorsi, di progressione in carriera, di scelta obbligatoria immediata con una scadenza di qui a poco tra funzione requirente e funzione giudicante; materie, queste, per le quali ogni intervento può essere di pregiudizio grave e non riparabile. Si parla poi di un decreto attinente alla sfera disciplinare. Anche qui si comprende benissimo come, se entrano in vigore, come lo sono entrate, norme sbagliate o addirittura pericolose, venga attinta la sfera professionale e personale del magistrato, che da norme sbagliate o pericolose può ricevere danni gravissimi. Pensiamo, oltre che alla reputazione, alla sospensione dal servizio, al trasferimento, alla rimozione. È ovvio come esistano margini di discussione, come non tutte le norme entrate in vigore siano sbagliate. Da qui deriva la nostra dichiarata disponibilità al dialogo e al confronto. Il fatto è però che, nonostante siano pressoché pronte le nostre proposte di legge in materia, bisogna decidere nell'immediato per questa fase transitoria,

Non mi nascondo che, se il disegno di legge del Governo fosse rimasto nella sua formulazione originale, si sarebbero creati dei problemi proprio per la fase transitoria. Il Governo, però, è intervenuto sul punto con l'emendamento 4.0.600, che vuole introdurre l'articolo 4-*bis,* volto proprio a regolamentare il regime transitorio. Ora, che la scelta tecnica adottata non sia la migliore mi pare forse indubitabile. Di qui a parlare di mostruosità giuridica, però, ce ne corre, in quanto la formulazione letterale dell'articolo 4-*bis*, proposto dal Governo, è chiara e precisa: da una parte, il comma 2, secondo cui sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite nel vigore dei decreti legislativi che vogliamo ora sospendere; dall'altra, la parte iniziale dell'articolo, il comma 1, parla di un sistema di norme - che viene specificamente indicato - che continua ad applicarsi. Sono forse espressioni non felici, se vogliamo, ma molto chiare e, comunque, di facile interpretazione ed applicazione. In conclusione, ribadita la nostra volontà di lavorare assieme all'opposizione per far funzionare in maniera efficace ed efficiente il pianeta giustizia, anche attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario, ritengo comprensibile, logica ed inevitabile la nostra volontà di regolamentare da subito e con urgenza la fase transitoria,

perché avverto la necessità personale di lasciare agli atti la traccia di un dissenso rispetto alla proposta formulata dal Ministro della giustizia. Nessuno potrà mai, in quest'Aula, mettere in discussione la qualità e la fermezza dell'atteggiamento di forte opposizione che nella scorsa legislatura mettemmo in campo contro la proposta di riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dell'ex ministro Castelli e portata avanti con arroganza da tutta la Casa delle Libertà,

piegati alla necessità di mettere in campo una prova muscolare che servisse a ridurre l'indipendenza della magistratura e a limitare, attraverso il sistema incrociato dei concorsi e delle opzioni, la funzionalità dell'apparato per determinare forme subdole di acquiescenza. Abbiamo esultato di fronte al messaggio alle Camere del Capo dello Stato che richiamava il legislatore al rispetto di quei precetti costituzionali che sono il fondamento di uno Stato di diritto moderno e credibile, nella considerazione che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura costituiscono un patrimonio di garanzia complessivo del sistema che rappresenta un patrimonio comune a tutti i cittadini. Ma oggi, signor Presidente, rispetto alla reiterata proposta di generalizzata sospensione di tutti e tre i decreti legislativi al nostro esame, non posso non rilevare che l'atteggiamento del Governo si appalesa debole ed ingiustificato.

La correzione, l'intervento puntuale, signor Presidente, era la regola; la sospensione era l'eccezione. Adesso, invece, la sospensione incondizionata diventa la regola generalizzata da attuare, limitandosi alla sterile e ripetuta enunciazione delle eventuali modifiche da apportare non si sa quando, non si sa dove. Se questa è la foto realistica della situazione, preferisco non partecipare ad un'operazione che considero ingiusta ed inopportuna per il Paese. DIVELLA *(AN)*. Ma come? Quando si è deciso di tentare una prima regolamentazione delle professioni, si è scelta la strada del decreto-legge, scontrandosi con tutti gli ordini, ed ora che si potrebbe intervenire su almeno su almeno due dei tre decreti, ritoccandoli, che cosa facciamo? Ne sospendiamo l'efficacia e creiamo un sistema monco ed inapplicabile, ancor più permeato dall'incertezza e dalla precarietà. Sul punto, una prima preliminare considerazione s'impone: l'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge delega incide in modo di per sé irreversibile sulla disciplina previgente. La sospensione dell'efficacia di tali decreti - si ribadisce - una volta che sono tutti già entrati in vigore non comporta alcuna automatica reviviscenza delle disposizioni che regolavano la materia anteriormente alla riforma operata nella XIV legislatura. È questo un punto che deve essere essere affrontato, perché determinerà una situazione di incertezza che il Paese non merita. Ma andiamo per gradi. Nella relazione che accompagna il cosiddetto disegno di legge Mastella è scritto che la reale motivazione - riassumo - per cui occorre immediatamente procedere alla sospensione è che, diversamente, entreranno in vigore decreti attuativi che avrebbero bisogno di un organismo di gestione - il riferimento è al CSM - nel pieno delle sue funzioni e che invece troverebbero un CSM debilitato e probabilmente debilitato ancor più dal fatto che per l'elezione della componente laica chissà quanto tempo sarebbe stato è verificato esattamente il contrario. Il CSM è stato eletto immediatamente, anche la componente laica è stata immediatamente e in una sola votazione eletta a rappresentare interessi generali del Paese. E allora, la motivazione la motivazione della sospensione dove è? Se volessimo essere ancora più fiscali, nell'analisi tecnica normativa legata al decreto è specificato «la concreta operatività dei decreti dipende dall'operatività del Consiglio superiore della magistratura. Da ciò la necessità del presente intervento normativo volto a sospendere l'efficacia dei decreti legislativi sopraindicati, in modo che la loro operatività coincida con la costituzione dell'organo di autogoverno». Per rendere operativo il sistema occorre che l'operatività dei decreti legislativi coincida - lo dice il Governo - con la costituzione dell'organo di autogoverno. Allora, se queste sono le motivazioni che enuncia il Ministro, sottese al provvedimento, resto veramente perplesso, perché non riesco a rinvenire la necessità di questo tipo di intervento. Veniamo, allora, al merito. Appare incontestabile la complessità di un intervento correttivo in merito al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, perché tutta la parte relativa alle procedure concorsuali, alle opzioni e all'accesso rappresenta un autentico *vulnus*, insuperabile rispetto all'indipendenza della magistratura. Rispetto a questo decreto, quindi, riconosco - come ho già fatto in Commissione - che occorrerà riscriverlo tutto, non apparendo assolutamente condivisibile la scelta operata dalla precedente maggioranza. Questo per me è dunque l'unico decreto legislativo rispetto al quale il provvedimento di sospensione potrebbe trovare effettivamente una motivazione accettabile. Ma rispetto agli altri due? Rispetto al decreto n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione dell'ufficio della procura, o al decreto n. 109 del 2006, che reca la normativa sugli illeciti disciplinari, quali sono le reali motivazioni che ci hanno impedito un intervento puntuale? Non riesco a comprenderlo, comprenderlo, se è vero, come è vero, che già intervenendo in sede di illustrazione del suo programma di Governo lo stesso ministro Mastella si preoccupava di delimitare le correzioni e le modifiche che avremmo dovuto apportare. Non voglio leggere il Resoconto stenografico, ma ricordo a me stesso che, per quanto riguarda il decreto n. 106 del 2006, si ragionava del modello organizzativo che in qualche modo doveva essere considerato anche dal CSM e ci fu un coro quasi unanime che concordava con il Ministro, così come la previsione di revocare l'affidamento dell'incarico giudiziario dell'indagine al pubblico ministero non poteva che essere motivata e l'eventuale revoca non poteva che essere sottoposta al CSM. Tutti d'accordo. Allora, quattro mesi fa, fa, l'ho ribadito in Commissione e ora le proposte di modifica dove sono? Per quanto riguarda la normativa sugli illeciti disciplinari, già allora il ministro Mastella precisò, intervenendo in Commissione (ed era la prima uscita di questo Guardasigilli), che sicuramente occorreva intervenire sulla tipizzazione. Siamo perfettamente d'accordo. era il problema dell'obbligatorietà della azione disciplinare, che andava contemperata prevedendo la possibilità in capo al procuratore generale di disporre una forma di archiviazione. Eravamo e restiamo tutti d'accordo. Le proposte di modifica dove sono?

molti dei componenti della Commissione nell'ascoltarlo condividessero e io personalmente mi permisi di esprimere concretamente quella posizione. Tutto inutile. Così come inutilmente ho riproposto la mia posizione, anche intervenendo successivamente in Commissione nel merito del provvedimento. L'ordine - mi spiace dirlo - era di blindare ogni cosa, anche la possibilità di emendare nel merito, ricorrendo a un'interpretazione, che personalmente considero abnorme, di un articolo del nostro Regolamento. Rispetto a questo contesto, un parlamentare dell'Ulivo è libero di dire che non condivide tale impostazione, sì o no? È libero di dire che questa sembra essere una controriforma debole e pasticciata, che corre il rischio di produrre maggiori incertezze e precarietà? Posso ricordare a me stesso che molto spesso le sospensioni diventano rinvii *sine die*? Posso rammentare a me stesso che la prima proposta di regolamentazione del disciplinare dei magistrati è stata presentata dal ministro Darida, *anno domini* 1982 (eravamo nell'VIII legislatura), seguita dalla proposta di legge del ministro Martinazzoli nella IX, dal disegno di legge Vassalli nella X, riproposta dallo stesso Vassalli nell'XI, con un disegno di legge che venne approvato dalla Camera, ripresa ancora da Mancuso nella XII e da Flick nella XIII? Posso ricordare a me stesso che sono venticinque anni che discutiamo del disciplinare dei magistrati e non riusciamo ad approvare uno straccio di norma e del senatore Polledri)*. Lo posso ricordare a me stesso, rivendicando la capacità di rivisitare storicamente le Aule di questo Palazzo, che non possono parlare se non quando noi diamo loro voce, come in questo caso? È chiaro che il sospetto che viene a qualcuno, che su alcune materie sia meglio non intervenire, che non si possa intervenire, comincia a diventare un sospetto che si materializza e personalmente vorrei scacciare questo cattivo pensiero, ma penso che non sarà possibile. Posso ricordare a me stesso, ad esempio, che la Bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, nella XIII legislatura, propose un testo del novellato articolo 123 della Costituzione che iniziava prevedendo che «L'azione disciplinare è obbligatoria»? Perché allora sì e adesso ci spaventiamo della previsione di obbligatorietà dell'azione disciplinare? Non lo so, continuo a chiederlo. Posso ricordare a me stesso che la sentenza n. 52 del 1976 della Corte costituzionale prevede la compatibilità di modelli di organizzazione gerarchica delle procure, chiaramente ragionando sul modello di un'altra norma? Ed allora, considerando conclusivamente che il ministro Mastella è venuto a precisare in Aula, all'inizio di questa discussione, che le sue ipotesi di modifica per i decreti nn. 106 e 109 restano sostanzialmente le stesse che aveva già illustrato in Commissione, ritengo di non poter condividere una tale impostazione e manifesterò il mio dissenso in modo chiaro e leale, avendo già ribadito - e tengo a precisarlo - tale mia posizione sia al Gruppo, sia al Presidente del Senato. Dissenso che esprimo - lo voglio dire chiaramente, in conclusione - anche rispetto alla proposta di strani organismi paralleli (Comitati ristretti tra maggioranza e opposizione) che dovrebbero riunirsi non si capisce come e dove, che offendono le istituzioni parlamentari che prevedono le Aule delle Commissioni e delle Camere per affrontare i percorsi legislativi. Le leggi si fanno in Parlamento: vi chiedo di non rinunciare a discutere, vi chiedo di poter esprimere chiaramente la mia posizione critica. *(Applausi

avviene oggi nelle procure, come abbiamo ascoltato, e il capo dei Lanzichenecchi, probabilmente, è tale ministro Castelli. Infatti, molti giudici, signor Presidente, sono approdati in quest'Aula e propongo di considerarli rifugiati politici,

clima apocalittico viene probabilmente smentito. Siamo nel Paese dei paradossi. Abbiamo affrontato quest'estate l'emergenza nelle carceri con una velocità invidiabile, come provvedimento legislativo: l'indulto. l'indulto. Forse qualche giudice poteva alzarsi e ricordare il lavoro dei giudici e la loro professionalità, tutto quel lavoro svolto (istruttorie e quant'altro) che in qualche modo veniva sicuramente messo da parte. Ora, però, che dobbiamo dare una risposta ad una categoria, anzi ad un intero settore, quello della giustizia, che non comprende solamente i magistrati, contenti di questo provvedimento, ma anche gli avvocati, scontenti come abbiamo sentito poc'anzi, i cancellieri, gli operatori e - ricordiamo - anche i cittadini, cosa rispondiamo? l'efficacia delle disposizioni è sospesa fino al luglio 2007, come abbiamo ascoltato. E nel mentre? La giustizia, continua a zoppicare, i cittadini non ottengono la certezza del diritto e, insomma, tiriamo a campare anche con questo provvedimento.

noi rimandiamo questo fino al luglio 2007. Si dice che occorre la riorganizzazione di interi settori dell'apparato giudiziario. Bene, perché non farla oggi? Rinviamo l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, come abbiamo sentito poc'anzi. La disciplina delle relative sanzioni, della procedura per la loro applicabilità, nonché la modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati? Rinviata. La nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché la materia della progressione economica e di funzione dei magistrati? Rinviata. Certo, a qualcuno fanno comodo questi rinvii. E' una cambiale che questa maggioranza paga all'Associazione nazionale magistrati. E' vero e reale quello che dice anche l'ex presidente Cossiga. Chi invece vuole accedere alla magistratura e svolgere il proprio lavoro con onestà, senso del dovere e rispetto dei princìpi costituzionali dovrà aspettare. Dobbiamo essere onesti, con noi stessi prima di tutto e, nel limite del possibile, sgomberare il campo dall'ipocrisia. La *lobby* dei magistrati - ci consentano di chiamarla come tale - esiste, lo sappiamo, e non ha assolutamente piacere che si intervenga con nuove regole trasparenti, legate all'efficienza e alla produttività, con meccanismi che vanno a premiare giudici onesti, professionisti (e siamo convinti che siano la maggioranza),

è dunque il vero punto di partenza? Cosa chiede il cittadino allo Stato in materia di giustizia? Processi in tempo ragionevole; giudici competenti, autonomi, indipendenti,

la valutazione psichiatrica la fa chi ha il brevetto per le caldaie, la fanno i cacciatori, i vigili del fuoco e altri ancora. Pensiamo

Senza pensare poi ai rapporti con gli organi di informazione. La riorganizzazione delle procure segue la linea di un miglioramento fondamentale della giustizia in uno dei suoi aspetti fondamentali, con il procuratore capo unico titolare dell'azione penale e unico a poter avere rapporti diretti con i *mass media*. Eviteremmo, a mio giudizio, quelle esternazioni che in questi anni hanno invelenito il clima politico del Paese.

anche e soprattutto di qualcuno di sinistra) farà sì che presto faranno carriera i migliori magistrati in circolazione, con particolare riferimento alle giovani leve, e questo non potrà che far bene alla giustizia. La sinistra di tutto questo cosa vuol fare? Rinvia.

Rimane un ultimo aspetto: il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti. Da più parti viene detto che una separazione delle carriere non è di per sé segno di mancanza di democrazia e autonomia della magistratura. Allora, a giudizio della Lega Nord, occorre non rinviarla, ma rinforzarla e iniziare un nuovo e stimolante *iter* per tutti. La formazione dei giudici e dei pubblici ministeri oggi, nel 2006, deve essere diversa, perché i compiti sono diversi, così come la loro inclinazione professionale. Chi ha avuto compiti di indagine non può trovarsi in un attimo a passare a competenze giudicanti e viceversa. Dobbiamo abbandonare la difesa dei benefici dello *status* *quo*. PRESIDENTE.

e di molte cose abbiamo già ragionato anche in Commissione. Come Gruppo di Rifondazione Comunista siamo favorevolissimi alla sospensione, proprio perché i tre decreti e tutta la riforma dell'ordinamento giudiziario del centro‑destra avevano scardinato l'impianto costituzionale che in questo nostro Paese e con questa Costituzione democratica costruiva una figura di giudice liberale terzo e indipendente, ovviamente speculare e anzi strumentale al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Pertanto, non si poteva rispettare il principio di uguaglianza in assenza di un giudice terzo soggetto anch'esso alla legge e non alla gerarchia, soggetto a un a un regime indipendente, strumentale anche proprio alla sua indipendenza. Quindi, l'indipendenza del corpo giudiziario come garanzia anche dell'indipendenza del singolo giudice. Un giudice che non essendo soggetto alla gerarchia potesse giudicare secondo legge, realizzando quel principio che abbiamo più volte definito del potere diffuso.

avevano nelle ideologie dell'epoca. Uscivamo da una dittatura molto feroce e quindi si voleva un giudice non soggetto

Ma il Costituente non aveva nemmeno come punto di riferimento un giudice ideologizzato che potesse rispondere ad un'idea di sinistra, perché allora legalità della sinistra, almeno in campo internazionale, era quella di una legalità socialista che aveva

di una riforma organica dell'ordinamento giudiziario che certamente può salvare anche alcune parti della riforma Castelli.

dovrebbe essere attento ad essere, ad apparire, che dovrebbe stare attento ad essere equilibrato e tanti altri aggettivi per i quali scatterebbero ipotesi disciplinari e a causa dei quali un giudice molto accorto potrebbe solo scegliere il percorso da casa all'ufficio e dall'ufficio a casa, proprio per evitare drammi ulteriori. dubbio, comunque, che una volta stabilito un codice rigido, tipicizzato, l'azione disciplinare deve essere obbligatoria: ci sarebbe una illogicità tra una disciplina rigida

un potere di archiviazione per le denunce infondate. Questo è tanto più facile quanto più ci sia una tipicizzazione vera.

si imponga una rigida distinzione delle funzioni. Certo, la riforma Castelli impedisce qualsiasi vera osmosi tra giudicante e requirente; però, non vi è dubbio che non si può neanche consentire il caos attuale per cui il giudizio di professionalità per il passaggio da una funzione all'altra è quasi sempre basato sulla sulla carriera, sull'età del magistrato che aspira ad un'altra posizione. E non vi è dubbio che non è plausibile

ci distingue, questo sì, dagli altri ordinamenti giudiziari. Quindi, una rigida distinzione, con un passaggio che deve essere motivato non attraverso questi esami e questa farraginosità, ma attraverso un esame serio ed una valutazione seria da parte del CSM. Tali funzioni, inoltre, vanno esercitate in altro distretto,

non c'è dubbio, infatti, che in alcuni Paesi la giustizia funzioni meglio, però dobbiamo storicizzare l'ordinamento giudiziario del nostro Paese,

ma abbia di mira soprattutto i diritti dei cittadini.

In effetti, la giustizia diventa ancora terreno di scontro e questa volta - lo dobbiamo riconoscere - per esclusiva responsabilità della maggioranza che ha scelto la strada dell'estremizzazione. invocare la sospensione di leggi vigenti nel nostro Paese con lo scenario dei conflitti intertemporali che sono dietro l'angolo - e che non sono assolutamente facili - significa determinare un'obiettiva situazione di scontro. La giustizia, l'ho detto tante volte, è terreno sul quale le convergenze dovrebbero essere

considerando l'analogo atteggiamento da lui avuto in occasione del decreto Bersani - quei soldati di Franceschiello che facevano la faccia feroce, ma poi si glorificavano in ritirate maestose. Vorrei sapere se alle parole trucide che egli ha dedicato alla maggioranza alla quale organicamente appartiene, parlando di progetto debole e non giustificato, farà seguire un atteggiamento coerente con la dichiarazione di voto.

sopravvissuta, nonostante la transitorietà delle norme, al 1948 - anno di entrata vigore della Costituzione repubblicana - al 1955 - anno di insediamento della Corte costituzionale - e all'alluvione delle leggi che si ponevano, naturalmente, in contrasto logico con quell'apparato normativo, che risentiva di una concezione dello Stato in cui

non c'è stata mai nessuna volontà di decentrare queste attività minori del Consiglio superiore della magistratura. Se oggi un magistrato si trova a dover chiedere un giorno di malattia, lo può fare, ma la sua

che è l'articolo filtro in base al quale il Consiglio superiore della magistratura, sulla base del parere dei consigli giudiziari, deve determinare la capacità e la possibilità di un magistrato di passare dalla funzione giudicante a quella requirente - si renderebbe conto che si è trattato di un passaggio automatico e deresponsabilizzato. Questa è la verità: tali prassi distorsive hanno creato, qualche volta anche in maniera aggressivamente tumorale, il potere della magistratura delle correnti, che ha finito per parlamentarizzare il Consiglio superiore della magistratura.

delle istituzioni, è stato trasferito all'interno del Consiglio superiore della magistratura, che è diventato l'arbitro non solo della vita dei magistrati, ma della vita della politica giudiziaria del nostro Paese. Questo è un dato di fatto.

perché sia il Ministro, sia l'Associazione nazionale magistrati, sia Mancino, sono entrati in maniera pesante in questo dibattito e per certi versi lo hanno condizionato o tendono a condizionarlo. Il Ministro ha giocato di fioretto perché è venuto qui, è stato volatile ed ubiquo, saltellante ed ecumenico, perché ha detto tutto e il contrario di tutto

Le obiezioni sono venute, a cominciare da quella del senatore Valentino (che ha parlato all'inizio della seduta); avremmo potuto incontrarci prima, come hanno detto tutti e come continuiamo a dire ancora adesso. Ma, di fronte ad un problema importante come quello della giustizia, ogni marginalità temporale può essere sfruttata e quindi noi ci auguriamo, per quelle voci che aleggiano nei corridoi e che si sentono anche in quest'Aula così vuota ma così significativamente piena di contenuti e di concetti, che domani mattina,

in questi mesi, che tradizionalmente noi giuristi di provincia definiamo diritti quesiti, e che creeranno gravissimi problemi, che hanno creato già discriminazioni,

passione politica. Noi ci auguriamo che ciò non sia e che domani possa esserci uno spiraglio di discussione e di dibattito più ampio. Ho sentito tuonare contro l'Associazione nazionale magistrati.

perché l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza dei magistrati sono un bene di ogni società civile e di ogni democrazia. Siamo noi ad esigere che nei magistrati prevalga l'autonomia, l'indipendenza e l'imparzialità, senza quelle distinzioni celestiali fra imparzialità apparente e imparzialità sostanziale, perché l'imparzialità è una e basta: non esistono queste distinzioni; l'ho potuto verificare e sperimentare proprio presiedendo la sezione disciplinare Non mi scandalizzo che l'Associazione nazionale magistrati rivendichi un ruolo di interlocuzione, perché è un soggetto né indifferente, né neutrale: non dev'essere un soggetto belligerante,

L'ultimo documento approvato l'altro ieri dall'Associazione nazionale magistrati e l'ultima dichiarazione che Giuseppe Gennaro, presidente della stessa, ha reso tracciano però simbolicamente una linea temporale gotica invalicabile: se entro il 28 ottobre non dovesse passare questa legge, loro sarebbero costretti allo sciopero.

stabilire date così ferme e fare affermazioni di questo genere mi sembra sia un metodo che non possa e non debba essere condiviso. Qual è il problema? Ho sentito prima - credo fosse il collega Casson - far riferimento

Sì, forse molti concorsi non servono, lo riconosco con molta onestà ed obiettività. Ma perché si è arrivati a questo? Voglio dirlo con grande sincerità. Non condivido quanto l'attuale componente del Consiglio superiore della magistratura, ed abituale notista de «l'Unità», il consigliere Livio Pepino, scrive da tempo, ossia che questa riforma vorrebbe determinare giudici su misura ed omogenei. A mio parere, gli unici giudici omogenei che ho conosciuto nel corso della mia esperienza diretta, sono quelli che escono dal sistema delle valutazioni di professionalità del vecchio Consiglio superiore della magistratura. Su questo punto siamo tutti d'accordo, perché, se parlo singolarmente con i magistrati, loro si dichiarano d'accordo con me: me: sono state queste prassi distorsive - lo ripeto ancora - a determinare una situazione tale da far ritenere che soltanto l'omogeneizzazione esclusivista e corporativa dei magistrati possa e debba essere premiata.

anni. Dobbiamo porci invece nel filone e nell'alveo delle grandi scuole di formazione dei pubblici dipendenti e dei magistrati, come in Francia con la scuola di Bordeaux, la *Grande École* della pubblica amministrazione francese. il Paese va avanti, ma se continuiamo ad avere il respiro corto del circolo vizioso delle appartenenze, non potremo determinare condizioni di miglioramento. In

sulla scia dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, approvata in Europa, determinava. Avanzo pertanto il seguente ragionamento: dal 1980 al 2000 i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati sono stati meno di 1.800.

anche se così dovesse essere, la legge attuale ci dà la possibilità, con interventi additivi che provengono dall'interpretazione corretta delle decisioni della Corte costituzionale, di creare più sezioni disciplinari all'interno dello stesso Consiglio superiore della magistratura.

debba essere mantenuto nel nostro ordinamento? Perché determina le condizioni di eguaglianza fra i cittadini. I magistrati che non voglio essere considerati cittadini dimezzati debbono ritenersi cittadini come gli altri. Questa è una norma di civiltà che deve entrare immediatamente in vigore e vi sono rimedi per porvi riparo. Sono convinto che, perlomeno sotto questo profilo, la battaglia sia perfettamente giusta. Mi spiace che non siano presenti i senatori a vita,

Qui c'entrano sia l'etica che l'estetica nell'opporsi ad un disegno di legge che vuole stabilire princìpi di uguaglianza e di civiltà. Queste sono le ragioni sulle quali cresce il motivato dissenso mio e di Alleanza Nazionale.

nel Paese, durante la campagna elettorale e in tutte le occasioni, ne veniva preannunciata la cancellazione rapida, immediata, come primo atto della legislatura successiva, qualora il fronte opposto avesse vinto le elezioni. E questo la dice lunga sul significato reale

durante l'esame di questo disegno di legge, hanno sentito il bisogno di ribadire che non si trattava di spazzare via una riforma dell'ordinamento approvata nella precedente legislatura e da altra maggioranza,

Il dibattito ha messo purtroppo in evidenza che, se dovesse restare tale ed essere approvato il disegno di legge sulla sospensione, si determinerebbe di fatto la cancellazione di un provvedimento importante, importante, approvato nella precedente legislatura. Questo è già un fatto gravissimo per la democrazia italiana e per il significato che assume il Parlamento nella democrazia italiana.

democrazia, ritengo che concepire l'alternanza e il bipolarismo come la cancellazione di tutto ciò che è stato fatto nei cinque anni precedenti sia forse la cosa più grave che si possa immaginare per distruggere la democrazia. Figuratevi che cosa è e che cosa può essere di un Paese quando le energie politiche sono destinate alternativamente a distruggere tutto ciò che è stato fatto prima.

aveva dichiarato, durante tutto l'*iter* della precedente approvazione della legge, la sua aperta contrarietà, ma non poteva e non doveva ipotizzare la cancellazione di una legge dello Stato,

pessimismo mi sembrò quasi allontanato dall'intervento che il ministro Mastella fece all'inizio di questa discussione, quando riprese la parola dopo la sua iniziale relazione; infatti, nel discorso del Ministro stranamente comparvero una serie di considerazioni che erano punti di favore rispetto alla riforma precedente. Mastella in quest'Aula - ho riletto, così come aveva invitato

dell'attuale maggioranza: uno degli ultimi di quelli ascoltati è stato un discorso forse ancora più deciso di quanto sono stati quelli dell'attuale minoranza. Perché allora non si dà il via

che significa fatalmente voler cancellare la riforma perché nei termini previsti non è possibile, dopo aver compiuto un atto così grave nei confronti dell'attuale minoranza, pensare di riprendere il discorso sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, non non si dà il via a quello che tutti hanno dichiarato di voler fare e che l'attuale minoranza ha ripetuto in varie occasioni e in molti discorsi di questo dibattito? Perché non si deve sostanzialmente operare individuando quali sono i punti del dissenso e ragionare su di essi, per vedere in che misura la riforma dell'ordinamento giudiziario può essere corretta? Avrei capito la posizione dell'attuale maggioranza se vi fosse stato da parte della minoranza, cioè da parte nostra, un arroccarsi su una legge varata dopo due anni di dibattito,

a mio avviso, è un gravissimo atto contro la democrazia e verso la possibilità di avere finalmente una riforma dell'ordinamento giudiziario con quel tipo di partecipazione che il Presidente della Repubblica ha ripetutamente richiesto.

non imbrogliamo gli italiani; almeno non imbrogliate - e lo dico alla maggioranza - gli italiani, ma dite la verità: se volete cancellare la riforma è perché siete eterogestiti e perché ritenete di esservi impegnati in tale direzione. Ditelo: se ce la fate, cancellate la riforma;

che era il momento di introdurre, dopo cinquant'anni di attesa, una legge sulla disciplinare che riguardasse i singoli casi, il principio di tassatività, l'obbligo dell'azione (princìpi, quasi tutti, riconosciuti da ogni parte politica), oggi ci si chiede di votare la sospensione di un punto che non trova nessun contrasto se non - da quanto mi risulta - con due o tre ipotesi (e per cambiarle sarebbe sufficiente, forse, un lavoro in Commissione o in Aula di qualche giorno, non di qualche mese o di qualche anno). In conclusione, voterò contro questa sospensione per un motivo molto semplice: è un modo indiretto, subdolo, bugiardo bugiardo di mettere da parte una riforma che tutti, a parole, avremmo voluto e dovremmo, invece, approvare Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, certamente l'ora tarda mi consiglia di essere molto conciso, anche se, debbo dire, almeno gli ultimi interventi che ho avuto occasione di ascoltare - li ho ascoltati quasi tutti, ma soprattutto gli ultimi richiedono una più attenta riflessione - anche per il prestigio delle persone che hanno parlato, meriterebbero risposte puntuali. Vorrei, allora, brevemente toccare alcuni punti. Nella scorsa legislatura, tutti quelli che erano presenti ricordano certamente che sull'ordinamento giudiziario si sono svolte lunghe discussioni, discussioni, anche aspre, e confronti duri. Desidero subito precisare che la riforma dell'ordinamento giudiziario non è stata una scelta governativa o una scelta

che la scelta dell'allora Ministro di affrontare questo problema merita apprezzamento. Poi come andò e come fu affrontato è altra ma risolvere il problema dell'ordinamento giudiziario era un dovere. È una grave responsabilità del Parlamento - ho avuto occasione di dirlo più volte - non aver affrontato un tema fondamentale e causa, forse non ultima, della crisi della giustizia nel nostro Paese. La VII Disposizione transitoria della nostra Carta costituzionale dice in modo chiarissimo che l'ordinamento Grandi del 1941 è incostituzionale: dev'essere cancellato e riscritto secondo il modello voluto dalla nostra Costituzione. Non si è fatto nulla. Eppure, se guardiamo al sistema giudiziario, nell'attuale ordinamento, ci accorgiamo che esso è radicalmente mutato rispetto ad allora. Vi sono giudici che sono scomparsi, come il giudice istruttore, e vi sono giudici nuovi, come il Gip e il Gup. Che cosa è successo in effetti? È successo che in parte il Parlamento, in parte la Corte costituzionale, in parte la Corte di cassazione, ma soprattutto il Consiglio superiore della magistratura, con le sue circolari, hanno radicalmente mutato il sistema ordinamentale della magistratura. Condivido molte delle scelte fatte, ma non condivido che l'ordinamento giudiziario sia stato riformato attraverso le circolari del Consiglio superiore della magistratura. Non era questo

rispetto alle scelte che il Governo fece in quelle occasioni. Collega Ziccone, tutti vogliamo questa riforma, infatti abbiamo sostenuto con forza la necessità che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura poggiassero sul rafforzamento dei poteri di controllo, per esempio del Consiglio superiore della magistratura, che non sono quelli che ha ora esposto il collega Nicola Buccico, che pure è stato lì; si tratta di controlli assolutamente inefficaci.

lei non dimentica che siete stati voi a diminuire il numero dei membri del Consiglio superiore della magistratura, indebolendolo ulteriormente. Queste sono gravi responsabilità politiche nella visione complessiva della riforma del sistema giudiziario.

Potrei aggiungere che le parti che vanno già bene - e lei lo sa meglio di tanti altri, collega Ziccone - sono quelle alle quali noi abbiamo cooperato, anzi sono frutto della nostra iniziativa, del nostro dibattito, del nostro contributo.

superiore della magistratura è stata un'idea di Elvio Fassone. Non condividevamo quel meccanismo di controllo della Corte di cassazione, ma intanto l'istituzione fu una nostra idea ed è un'idea che noi apprezzammo. se lei legge la storia - adesso la ripercorrerò brevemente - di quel provvedimento, si renderà conto di come, mentre si progrediva nella discussione, improvvisamente entravano in gioco considerazioni endoparlamentari,

Èquesto il punto: questa legge è stata frutto di urgenze determinate da eventi esterni al Parlamento stesso, che hanno portato ad alcuni vizi profondi. Non mi può dire che è stata attuata la separazione delle carriere o delle funzioni: né l'una, né l'altra. Voi avete portato avanti quanto più possibile, senza la riforma costituzionale, che era doverosa, una separazione

Avete operato una distinzione di funzioni fittizia, nella quale però vi sono momenti che sono assolutamente inaccettabili.

la necessità di riprendere il discorso, sospendendo per un momento gli effetti che ne possono derivare, senza mettere in discussione la necessità della separazione o della distinzione delle funzioni o delle carriere: lo discuteremo. Certo è che, nel momento in cui questa legge dovesse produrre i suoi effetti, oggi un giovane che dovesse superare il concorso e dovesse scegliere

Di qui la necessità di sospendere questi effetti e di ridiscutere. Non capisco. Forse avreste voluto che fosse tutto cancellato e si ricominciasse da capo? Oppure non è invece opportuno sospendere gli effetti e ridiscutere punto su punto quale parte far vivere e quale modificare? Mi sembra una scelta ragionevole. Se poi a questo aggiungiamo ciò che il Ministro ha detto, e cioè quali parti intende ridiscutere (e mi sembra che gran parte

e non provocare subito effetti, magari drammatici, per poi modificare questa legge con norme transitorie? Mi sembra una scelta assolutamente ragionevole. Mi lasci ricordare - purtroppo qui siamo rimasti soltanto quelli che vivemmo quella esperienza, ma dato che poi questo intervento andrà sulle carte e sarà letto, sarà bene ricordarla anche a coloro che ora sono assenti - che il ministro Castelli presentò in Senato il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario nel marzo 2002. Cominciammo la discussione anche se aspra, fu molto positiva e stavamo giungendo al termine di quella fase in Commissione quando improvvisamente tutto venne sospeso. I lavori della legge delega vennero sospesi d'improvviso, dopo mesi di lavoro, perché nel frattempo intervenne un fatto tutti sappiamo a cosa mi riferisco): un processo che si celebrava a Milano con un ricorso in Cassazione per il problema del cosiddetto legittimo sospetto e con la presentazione di una legge *ad hoc*, la cosiddetta legge Cirami.

fino a quando, il 7 marzo 2003, il Consiglio dei ministri varò un maxiemendamento di modifica radicale del testo originario della legge delega, soprattutto in tema di progressione di carriera, ridisegnata con criteri meritocratici e di separazione delle carriere. È impossibile non mettere in fila questi eventi

ma che sarebbe stata certo di gran lunga più positiva. Per questo non mi sento di attribuire al ministro Castelli tutta la responsabilità. Fu il Consiglio dei ministri che decise con forza la presentazione del maxiemendamento. Se così fosse, potremmo anche ridiscutere e valutare quello che accadde. Ma non è finita, anzi. Quando il testo giunge alla Camera dei deputati è un testo radicalmente modificato. Il disegno di legge è riscritto più volte, in Commissione e anche in Aula. Al termine, ancora una volta, è presentato un maxiemendamento sul quale il Governo chiede la fiducia. Nel giugno 2004, la Camera dei deputati vota un disegno di legge totalmente diverso rispetto a quello presentato dal ministro Castelli e da quello votato al Senato. Quindi, il disegno di legge n. 1296-B costituisce la quarta stesura della riforma dell'ordinamento giudiziario. Ognuna di tali stesure è stata radicalmente diversa dalla precedente e nulla è rimasto dell'elaborato originario. Quando arriva al Senato, il disegno di legge, che - ricordiamolo - era stato approvato con voto di fiducia e il Ministro aveva detto che era assolutamente inemendabile, viene modificato con un nuovo maxiemendamento redatto e presentato proprio da quel Governo che aveva chiesto ed ottenuto la fiducia. Il grado di confusione è straordinario. Ma non finisce qui. il maxiemendamento è presentato solamente pochi minuti prima della scadenza del termine prefissato, lasciando a noi dell'opposizione la notte come termine per redigere i nostri subemendamenti,

In sintesi, la situazione è questa: abbiamo quattro testi ogni volta uno diverso dall'altro e ciascuno dei quali mai discusso compiutamente in Parlamento. L'ultima versione è approvata con voto di fiducia alla Camera ed è emendata in Senato dallo stesso Governo che, non soddisfatto dell'immane confusione creata, corregge i suoi stessi emendamenti che modificavano quel testo sul quale aveva chiesto e ottenuto una fiducia evidentemente mal riposta. Questa è la storia di questa legge: una storia confusa, arruffata e nella quale il Parlamento si è trovato di fronte a improvvisi cambiamenti di scenario,

non fa queste cose. Il Parlamento, dunque, ha approvato così questa legge. Come consentire che essa rimanga quando è stata permeata ed intrisa di questi umori ragionevoli? Tali umori sono risposte astiose e come tutte le risposte astiose non hanno nulla a che fare con la ragionevolezza e con la giustizia. Presidente, ricordo ciò che Dante fa dire a Cacciaguida: «Sempre la confusion delle persone principio fu del mal della cittade». Ecco, il male della nostra città, del nostro Paese, del nostro Stato è appunto la confusione. Questa è una legge permeata

di ridiscutere la legge non cancellandola ma sospendendone gli effetti per poterla discutere, sia la via più ragionevole. Non facciamo maxiemendamenti, non la riscriviamo quattro volte, vediamo di discutere insieme quello che si potrà fare. A quale fine? Come dice Dante, quello appunto di evitare la confusione, il male maggiore che possa colpire il nostro Stato. Nell'interesse di chi? Non dei magistrati,

questo è il punto fondamentale. Il Ministro che ha osato varare una riforma contro il parere della magistratura va cancellato, la riforma va cancellata come elemento plastico per definire il potere della magistratura in materia di giustizia». Credo che qui nessuno possa erigersi a Marco Catone e francamente il ministro Castelli esagera nel paragonarsi a Cartagine; forse ad Albalonga, ma Cartagine era una minaccia molto più forte per la civiltà romana. Non c'è un potere dell'ANM su di noi e nessuno vuole colpire il ministro Castelli. Mi sembra che sia un'esagerazione ingiustificata. Vogliamo riscrivere una legge necessaria al Paese, dovuta per impegni costituzionali, una legge che sia più serena, più vicina agli interessi dei cittadini, e i magistrati, gli avvocati, l'ANM o chicchessia non hanno alcun potere per influire sul nostro intendimento, quello sovrano del Parlamento che lavora nell'interesse dei cittadini. Questo è ciò che vogliamo e speriamo di perseguire nel migliore dei modi.